al primo anno della facoltà di giurisprudenza ci insegnavano, come insegnano oggi, che la legge è la composizione di opposti interessi nella ricerca costante e meticolosa di questa composizione, si concreta la funzione parlamentare di maggioranza e opposizione.

accogliere alcune delle nostre critiche per poi dire che occorre trovare un accordo; se non ci muoviamo, tra chi Rispetto all'intervento del presidente Salvini - come si dice a Milano - "con il cuore in man", ho trovato fuori luogo l'intervento della mia amica De Petris che ha voluto ricordare a Salvini di dover rivolgere lo stesso appello a Orbán per le leggi in vigore in Ungheria. Dobbiamo Dobbiamo ragionare su quello che dobbiamo fare noi, perché veniamo meno a quella che è una regola della democrazia, del Parlamento. La prima questione, è possibile che non si debba discutere? Penso alla posizione del Partito Democratico in Commissione e non mi interessa stabilire la data, anche se è vero quanto detto dal presidente Ostellari. Il 28 aprile c'è stata la prima seduta, ma non ha importanza. importante un aspetto fondamentale: non si è consentita la possibilità di discutere; non ho avuto la possibilità di trovare quel clima che nella passata legislatura fu trovato

Quando si dice che l'istigazione a delinquere deve essere punita, significa non avere presente qual è l'organizzazione del nostro sistema penale. Mi meraviglia che alcuni di voi che sono giuristi, forse migliori di me, non si rendano conto del contrasto evidente tra l'articolo 115 del codice penale, che dice che nessun cittadino italiano

insieme il tentativo di correzione anche della legge Mancino, perché dobbiamo ragionare in termini di correttezza.

l'interpretazione non solo di un dato fatto, di una specifica previsione legislativa, applicandola al caso concreto. Non è così. Si tratta di una libertà di interpretazione che avverrà da una parte all'altra dell'Italia anche in modo diverso. Come fate, allora, a non rendervi conto

È questo che mi fa inquietare e che non riesco a comprendere. Io non sono capace di schierarmi a priori a destra o a sinistra, con la maggioranza o con l'opposizione solo per mettere una bandierina Io voglio raggiungere il risultato di una norma che sia idonea a garantire ai nostri cittadini una tutela per chi si trova nelle condizioni previste dal disegno di e nello stesso tempo una garanzia a tutti i cittadini di non essere coinvolti in una guerra di religione in un certo senso. Molti infatti non intervengono in quest'Aula forse perché hanno il timore di ritrovarsi tacciati di omofobia per aver detto qualcosa che non ha alcuna volontà di essere inquadrata in quella fattispecie. Io mi domando

non dovrebbe avere la condizionalità del segretario del Partito Democratico.

Occorre allora individuare le ragioni che sono alla base di un'azione politica che probabilmente è fatta soltanto per acquisire qualche consenso. A me non pare che sia una cosa che faccia acquisire consensi: basta pensare al voto di ieri sulle pregiudiziali. Spaccare il Paese, spaccare il Parlamento in due è una cosa non da grandi politici, ma da politicanti.

del disegno di legge in esame, perché ci saranno molte altre occasioni per farlo nei prossimi giorni. Richiamo i colleghi al rispetto della Costituzione in una forma estremamente specifica: proseguire su questo provvedimento ignorando quanto è stato fatto pervenire in un primo tempo dalla Segreteria di Stato della Santa Sede e più specificamente - poi dirò perché - da due Chiese titolari delle intese. Nel nostro Paese la questione

alla fine della Seconda guerra mondiale e l'Italia si è impegnata a tutelare la libertà religiosa per esplicita richiesta degli Stati Uniti d'America, che avevano e hanno a cuore questo tema. Infatti, la nostra Costituzione in diversi punti si occupa della questione della libertà religiosa: nell'articolo 3, che prevede che non vi sia alcuna discriminazione per ragioni religiose, tutte le religioni naturalmente;

il rispetto della Costituzione dovrebbe essere insito in tutte le leggi e questa non è una novità. Quante volte nelle questioni pregiudiziali e sospensive, da entrambe le parti, nelle varie fasi in cui ci si trova all'opposizione, vengono sollevati dubbi sull'incostituzionalità di certe parti. Ma qui vi è un fatto procedurale che non lascia scampo: l'articolo 7 della nostra Costituzione Costituzione prevede che i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica siano regolati dai Patti lateranensi, che, quando è stata scritta la Costituzione, erano i Patti del 1929, poi rinnovati nel 1984 e firmati per la Repubblica Italiana dal presidente del Consiglio Bettino Craxi e dalla sua controparte, il Segretario di Stato della Città del Vaticano.

La nota verbale consegnata il 17 giugno dalla Segreteria di Stato del Vaticano all'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede richiama precisamente questo: richiama l'articolo 2 dei Patti lateranensi, che prevede la libertà per la Chiesa di professare il suo magistero e per i singoli credenti di praticare la propria religione. Qui non abbiamo un letterale richiamo alla situazione in cui siamo, anche se la lettera della Segreteria di Stato mi sembra che lasci pochi dubbi. La laicità dello Stato qui non c'entra nulla. Non c'entra nulla, perché si tratta di rispettare un trattato; che poi questo trattato sia con la Santa Sede anziché con un altro Stato (la Bulgaria, l'Algeria o chissà quale) poco rileva. Bisogna rispettare i trattati, specialmente quando sono specificamente previsti dalla Costituzione. nella Costituzione c'è anche l'articolo 8. Giustamente, i Padri costituenti vollero regolare i rapporti con la Chiesa cattolica, per le note vicende che conosciamo sorte dal 1870 in poi. Ma, per questioni di libertà religiosa, che deve essere garantita a tutti, previdero l'articolo 8, e cioè le intese con le altre confessioni religiose. Bene, fra quelle ci sono le intese con ci sono le intese con la Chiesa apostolica in Italia e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, entrambe approvate dal Parlamento nel 2012

la terzultima è la sigla da parte della Repubblica italiana e della confessione religiosa interessata. Per la Repubblica italiana quella sigla fu messa dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Enrico Letta, nome che a qualcuno di voi specialmente dovrebbe ricordare qualche cosa. *(Applausi)*. E non ha firmato perché voleva fare quello, ma perché rappresentava la Repubblica italiana. La firma vera e propria, che avviene dopo una serie ulteriore di accertamenti, viene fatta dal Presidente del Consiglio, che all'epoca si chiamava Romano Prodi (altro nome che dovrebbe essere familiare a molti). Ma quella firma, di nuovo ovviamente, non l'ha messa lui come persona; sarebbe come se l'avesse posta qualunque altro dei Presidenti del Consiglio, come se l'avessero messa Mario Draghi, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Mario Monti o qualunque Capo del Governo, perché rappresentanti la Repubblica italiana come noi rappresentanti la Repubblica italiana. In entrambe quelle intese c'è un articolo che poi è stato approvato per legge (sono leggi previste direttamente dalla Costituzione), dove c'è scritto:

c'è scritto: «In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa apostolica in Italia» - oppure della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni in Italia lo Stato, verranno promosse, previamente in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso». Questo è un obbligo preciso, e non una facoltà. Non siamo qui in questo momento a giudicare se i rilievi fatti da dette chiese siano corretti o meno. Abbiamo una norma prevista dalla Costituzione che ci dice che previamente bisogna dare retta a queste domande. *(Applausi)*. Altrimenti vuol dire calpestare la Costituzione in una parte dove tutela la libertà religiosa. Poi starà al Governo *in primis* dire cosa deve fare; ma non si può semplicemente ignorare questo, perché altrimenti vuol dire mettere sotto i piedi la parola della Repubblica italiana, che tra l'altro è stata data da Romano Prodi e da Enrico Letta. Volete fare questo? Questa è una cosa molto grave. Al di là delle ragioni portate da queste due confessioni religiose, c'è un impegno preciso della Repubblica italiana. Se riesco, nel tempo che ho a disposizione vorrei precisare che queste due confessioni hanno tenuto entrambe a dire che sono pienamente d'accordo con la tutela dei diritti e dell'uguaglianza delle persone che si riconoscono come LGBT e sostengono i loro diritti. Ciò è scritto nel testo delle lettere formali inviate al Presidente del Consiglio, e viene ribadito. Peraltro, entrambe le confessioni religiose hanno subito, anche in Italia,

dopo si dovrà votare per vedere quale tipo di sospensione ci sarà. Faccio notare che, se non viene data risposta - tra l'altro il Governo stesso dovrebbe dare risposta, perché chi firma le intese è il capo del Governo;

stringata e breve. Nel deliberato chiediamo sostanzialmente di sospendere l'*iter* del provvedimento e di rinviarlo al 27 luglio, per dare tempo alla Commissione di verificare se si riesce a trovare un accordo politico, per una gestione ordinata del provvedimento. Ci sembra una richiesta assolutamente di buon senso, anche perché

per una legge di civiltà, che serve al Paese? È tutto qui il tema su cui dobbiamo ragionare ed è necessario che ci sia chiarezza e trasparenza al riguardo perché, a seconda di come vogliamo giocare la partita,

della Lega, da Forza Italia o da Fratelli d'Italia, ma autorevolissimi esponenti del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle hanno messo in dubbio la definizione di identità di genere, ponendo la questione del rischio di un utilizzo opportunistico dell'aspetto del genere

del vostro schieramento che hanno posto la questione. Quando si parlava dell'indeterminatezza delle norme penali, una collega del MoVimento 5 Stelle è intervenuta su questo tema

mancano requisiti di tassatività e determinatezza, mentre il cittadino deve sapere con certezza quali sono le condotte che possono comportare una sanzione penale. Non ci possono essere dubbi, non si può lasciare tutto alla discrezionalità del giudice.

arrivare a chissà quando - per lavorare in Commissione, fugare i dubbi, superare le criticità e arrivare a una soluzione buona per il Paese. Noi riteniamo che sia questa, ragionevolmente, la logica che tutti quanti la logica che tutti quanti dovrebbero perseguire. Non vorremmo che, nell'epoca del distanziamento sociale, si fossero prese le distanze anche dal buonsenso. Forse bisognerebbe ritrovare un po' di buon senso e un po' di intelligenza politica su queste tematiche, anche perché tutto tutto dipende - come ho detto - da come volete giocare la partita: se il modulo, lo schema è o la legge Zan così com'è o morte, copiando un po'

stanno legittimamente decidendo, con un applauso, di dare un segnale di assenso su un passaggio di un intervento di un altro collega senatore. Ieri sono stato reputato colpevole di aver fatto un applauso insieme ad altri colleghi del Gruppo a un passaggio dell'intervento del senatore Salvini. La senatrice Cirinnà ha reputato corretto riprendere tale applauso e rendermi oggetto di lapidazione *social*, perché naturalmente non si è limitata solo a riprendere l'intervento,

senza naturalmente dire che quella pregiudiziale è stata bocciata grazie ai nostri voti. Presidente, la prego di intervenire e chiedo anche alla senatrice Malpezzi di agire nei confronti della sua collega del Gruppo

e anche augurargli un cordiale benvenuto nel mio mondo. Chi si espone nel dibattito *social* è fatalmente, prima o poi, oggetto di linciaggio.

e alla violenza, nella quale vediamo emergere, in tutta la sua nitidezza, la doppia morale che caratterizza alcuni partiti presenti in questo augusto

da qualsiasi parte esso provenga, perché fa parte della dialettica politica manifestare, anche in forme - se posso usare questo termine - sceniche, il consenso nei riguardi di tesi espresse in Ma - sa com'è - qui viviamo nella «Fattoria degli animali», per cui alcuni applausi sono più applausi degli altri e qualche odio è più odio di altri. In particolare, la battaglia che stiamo personalmente combattendo come forza politica in quella Commissione è cercare di far capire che l'odio o comunque l'istigazione al linciaggio - se tale è, naturalmente, perché poi c'è anche da fare un discorso su quando questo fenomeno si caratterizzi è deprecabile sia che venga dalle orrende schiere conservatrici, oscurantiste e barbare da questa parte, sia che venga dall'illuminata ed eletta schiera dei difensori del progresso e della democrazia,

noi, diventerebbe più facile addivenire a una sintesi politica e anche passare sopra, con buon senso, a incidenti che ci possono essere. Ma l'incidente diventa inaccettabile se viene da parte di quelli che si autoproclamano buoni, essendosi dimenticati la canzone di Gaber con la quale hanno convissuto nella loro ormai lontana giovinezza, e quindi una certa dimenticanza ci sta. La dittatura dei buoni non ci piace. Non ci piace nessuna dittatura, quella dei buoni ancora di meno, perché è particolarmente insidiosa e pericolosa, dal momento che si presenta lastricata di buone intenzioni, come deve essere ogni via di ogni inferno, che è in terra prima di essere nella vita che ci attende.

Sappiamo benissimo che tale divieto è scarsamente rispettato. Ho avuto però modo di verificare direttamente il filmato che è stato richiamato dal senatore Faraone l'angolo di inquadratura da cui è stata svolta quella ripresa non pone il dubbio che la stessa sia stata fatta dall'interno dell'Aula e da una certa ala dell'Emiciclo e non sicuramente dall'alto o, eventualmente, dalla stampa. Io sono abituato, purtroppo, a vedere che non c'è un divieto che viene rispettato se non esiste una sanzione. Quindi, essendo stato indicato un responsabile da parte del senatore Faraone, cui va la mia totale solidarietà, io chiedo che vi sia, da parte della Presidenza, un richiamo nei confronti dell'interessato,

io la ringrazio di questo suggerimento. Avevo già detto che avrei fatto svolgere l'indagine. Quindi, la ringrazio per avermi aiutato in questo lavoro. Ribadisco che la

non parlerò di questioni di Regolamento, che pure sono utili, ma non posso non partire dalla vicenda denunciata dal collega Faraone.

che la nostra eccezione di incostituzionalità, con la quale sostenevamo che il provvedimento in esame viola i sacri principi della Costituzione, è passata grazie ai voti del suo Gruppo, perché sono mancati solo 12 voti. È storicamente vero che voi avete votato contro la nostra eccezione di incostituzionalità. Collega Faraone, errare è umano, ma perseverare è diabolico. Fra poco si vota di nuovo. Dopo quello che è successo, ve la sentite davvero di sottolineare con un voto contrario

è piena. Ce ne sono tante! Non tante da poter determinare una maggioranza, ma ce ne sono tante che non accettano che qualcuno pensi in maniera diversa da come loro ritengono sia giusto pensare

violenza e una nuova cultura, che è figlia dell'intolleranza, che è figlia dell'odio, che è figlia della divisione e della discriminazione. *(Applausi)*. Voi state discriminando chi non la pensa come voi.

Non auguro a nessuno queste forme di discriminazione. Amici dei 5 Stelle, che siete giovani alla politica, fidatevi: non ce l'ho con voi, anche se certi atteggiamenti di alcuni di voi mi fanno veramente sorridere, e ripeto veramente sorridere. Non Non c'è più bisogno di dire che cosa potrebbe succedere se questo provvedimento dovesse passare a uno che sostiene semplicemente che è sbagliato che un transessuale, nato uomo - gareggi alle Olimpiadi con le donne. Uno può non essere d'accordo; ma, se io non sono d'accordo, non è un'opinione, diventa un reato. Ancora più grave è poi se dico - e rischio quattro anni di carcere, perché faccio parte di un movimento politico che lo sostiene dalla A alla Z - che un bambino non può essere adottato da una coppia di genitori dello stesso sesso. Non può essere però omofobia, visto che il responsabile di un organismo degli omosessuali di destra, che esiste, ieri, in un'intervista su tutti i giornali, ha stigmatizzato questa legge e queste forme di discriminazione. Noi siamo diventati, nostro malgrado, i vessilliferi della tolleranza, i vessilliferi di chi accetta il confronto, di chi vuole sapere come la pensi e non ha paura se uno la pensa diversamente. Questo è il dato per cui oggi siamo a favore delle questioni sospensive presentate non

avete immaginato di non andare a votare, perché il voto, come le opinioni, per voi è il massimo della paura.

colleghi, un momento di silenzio.

il Consiglio di Presidenza a prendere in considerazione l'adozione di un atteggiamento da tenere sempre e comunque rispetto a una serie di comportamenti assunti

per comportamenti rispetto ai quali avevo chiesto di intervenire con visione di filmati e individuazione di responsabilità. Vorrei citare, per tutti, il caso di un commesso che ha fatto una serie di evoluzioni sui banchi, certamente non per suo spirito acrobatico

Credo che, a quel punto, si potrebbe intervenire su molteplici aspetti, che personalmente censuro

Propongo pertanto che si tenga un Consiglio di Presidenza per valutare d'ora in poi qual è l'atteggiamento da tenere sempre, come interveniamo e come informiamo - non ce ne sarebbe bisogno - i colleghi su come ci regoleremo

tutte quelle aggressioni e istigazioni alla violenza che avvengono da parte di rappresentanti (consiglieri comunali, consiglieri regionali e così via), che non solo prendono posizione su alcuni aspetti, ma incitano all'odio e hanno degli atteggiamenti decisamente violenti. Sono dell'idea che lo spazio della politica, proprio perché è uno spazio di cui rivendico l'autonomia, di cui rivendico l'autonomia, indipendentemente da interventi delle autorità a vario titolo, debba intervenire incisivamente con provvedimenti molto chiari e molto severi. Questo farebbe sicuramente bene a tutti. bene a tutti. Concludo, signora Presidente, non volendo abusare della cortesia che mi ha accordato. Noto un avvicinamento, diciamo così, al diritto mite

da parte della Lega, e questo ovviamente non può che essere salutato con grande soddisfazione e grande gioia. Avremo per esempio occasione di riparlarne sulla riforma del diritto penale, sulle pene alternative, sui lavori di pubblica utilità e su una serie di questioni alle quali siamo certi che la Lega, mentre raccoglie le firme per il *referendum*, sarà sicuramente molto sensibile e attenta.

hanno avuto il compito di verificare i singoli comportamenti. Anche perché c'è un principio che va sempre rispettato, che a lei non sfugge, rispetto a quello che si afferma in Aula. La verifica serve proprio per appurare *si* *vera sunt exposita*. Quindi, daremo luogo a tutti gli accertamenti del caso.

come oggi, mi sembra di vedere in quest'Aula il tentativo, da parte di alcune forze politiche - per carità, legittimo - di raccontare una storia che non è così anche non soffermandosi sugli articoli del disegno di legge per il quale ieri chiedevano la pregiudiziale di costituzionalità e oggi la sospensiva, con le diverse formule che sono state presentate. Dico questo perché sembra davvero che ci siamo trasformati tutti in donne e uomini di buona volontà, tutti desiderosi di trovare una mediazione, tranne, molto probabilmente, le forze che hanno

alle forze che oggi dicono che c'è bisogno di più tempo, e che non si sono accorte che di questo tempo avevamo bisogno già negli otto mesi precedenti e che i nostri appelli alla possibilità di lavorare in Commissione sono tutti caduti nel vuoto, salvo poi accorgersi - dopo la spinta alla calendarizzazione - che forse la necessità di affrontare il disegno di legge c'era. Eppure, non se n'erano accorti prima, quindi solo da una settimana sta avanzando la narrazione di una volontà di portare a casa la legge. Mi chiedo, però, se ci sia stata la volontà di leggere il testo e se

è stato chiamato emendamento salva idee, voluto da tutto il centrodestra, votato all'unanimità, e posto come condizione per poter votare quell'articolo all'unanimità.

Avete cambiato idea, ma sappiate che quella norma è figlia vostra, la avete voluta, e a noi oggettivamente oggi il vostro sembra un pretesto.

per segnalare - in riferimento all'articolo 7 - una richiesta che il senatore Salvini ha avanzato ieri sera. Leggo dallo stenografico, Presidente. Nel suo intervento il senatore Salvini dice «Togliamo i bambini e togliamo l'educazione affidata alle scuole elementari: lasciamo alla mamma e al papà il diritto e il dovere di educare i propri bambini, non allo Stato».

l'articolo 7 del disegno di legge - non vorrei mai essermi confusa - che riguarda questa parte al comma 3, perché penso che il senatore Salvini si riferisse a questo nel suo intervento. Cosa dice il comma 3? che «In occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,

Presidente, la mia difficoltà è comprendere come possano loro non essere d'accordo con un'iniziativa che è contenuta all'interno di una legge che recita così, né più né meno, perché il riferimento è chiaro. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche che sono già indicate addirittura in una legge precedente. Si aggiunge però al comma 3, che prima ho letto e che spaventa così tanto, che il tutto deve essere legato al patto di corresponsabilità. Cosa dice il patto di corresponsabilità? Ve lo dico, colleghi, perché siete genitori, vi riguarda e dovreste saperlo. «Le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell'offerta formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie». Che cosa dice sostanzialmente? Quello che è già in vigore, che i genitori sono parte del processo educativo che non vengono tagliati fuori, che le scuole decidono insieme ai genitori, Presidente, - e qui chiedo aiuto al mio collega e amico Davide Faraone sulla base di un comma di una legge che già nel 2015 - quando la votammo e devo dire che con Davide Faraone, all'epoca sottosegretario all'istruzione, ci avevamo lavorato tanto

Signor Presidente, è giusto che si sappia perché il senatore Pillon dalla comunicazione non verbale che ha espresso ha dimostrato che davvero loro sono convinti che dal 2015 nella scuola sia stata introdotta una ideologia *gender*, che non esiste. Mi chiedo per quale motivo, per esempio, non abbiano mai proposto di abrogare quel comma. *(Applausi)*. Segnalo, però, Presidente, che grazie al lavoro

che indicano proprio le modalità cui le scuole si devono attenere nella lotta contro tutte le discriminazioni e le forme d'odio. di legge Zan si rifà a quello, né più né meno. Voi capite, quindi, che nel momento in cui ci dite che dobbiamo sospendere i lavori per trovare mediazioni su punti che però state narrando in maniera non corretta, un problema sulla chiarezza del vostro comportamento o quantomeno sulla sua buona fede lasciate che ci venga

non sono in gioco le buone maniere, è una questione interamente politica. Cercherò quindi di spiegare il motivo di questa mia affermazione. Una delle obiezioni al disegno di legge Zan riguarda il concetto di identità di genere, perché esso sarebbe estraneo all'ordinamento e comunque non sufficientemente chiaro, ma non è così. L'espressione è presente nella direttiva sull'attribuzione della qualifica di rifugiato, che richiama l'identità di genere tra i motivi di persecuzione; se ne trova menzione nella direttiva in materia di diritti di assistenza e protezione delle vittime di reato, ove si considera la violenza contro una persona a causa, tra l'altro, della sua identità di genere. L'identità di genere è presente nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione di Istanbul del 2011. Inoltre, nell'ordinamento penitenziario si enuncia il divieto di discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale. Quanto alla giurisprudenza, sin dal 1985 la Corte costituzionale ha riconosciuto un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, in base a cui acquistano rilievo l'insieme di fattori psicologici e sociali che contribuiscono a determinare una concezione del sesso come dato complesso della personalità. costituzionale del 2017), elemento costitutivo del diritto all'identità personale rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona, è stato ribadito dalla Consulta nel 2017 come aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registi anagrafici al momento della nascita con quello soggettivamente percepito e vissuto. Questa, che è la definizione del disegno di legge Zan, è tratta da una pronuncia della Corte costituzionale del 2017 Passiamo poi all'altra questione. Si dice che il disegno di legge Zan è inutile, perché le disposizioni per punire comportamenti violenti o discriminatori già esistono. È vero, perché è ovvio che pestare a sangue una coppia di omosessuali, come purtroppo è tragicamente avvenuto troppe volte nel nostro Paese, è già reato. Tuttavia il disegno di legge Zan non tratta di questo, ma di chi istiga a commettere tali reati. Per questo, e solo in questo senso, il disegno di legge Zan punta ad una attività educativa da svolgere anche nelle scuole per prevenire le discriminazioni. Stiamo parlando di istigazione al reato e l'attività formativa deve farne capire la gravità, ma è indubbio che ma è indubbio che il legislatore debba intervenire di fronte a un fenomeno che, proprio in assenza di specifiche fattispecie di reato, è statisticamente sottostimato, specialmente data la fortissima presenza che c'è sui *social network.* Per tutti coloro che sono contrari al disegno di legge Zan, il testo è ideologico, lesivo della libertà di espressione garantita dall'articolo 21 della Costituzione, perché non definisce con la determinatezza propria della legge penale quali siano gli atti discriminatori e, di conseguenza, quali opinioni vadano considerate reato perché idonee a determinare il concreto pericolo di un loro compimento. Anche questa è una clamorosa falsità. Innanzitutto il disegno di legge Zan non introduce una nuova fattispecie di reato, piuttosto estende i delitti già previsti contro l'eguaglianza, aggiungendo alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi quelle fondate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità. Quindi, quanti sostengono che si tratti di una proposta di legge repressiva della libertà di espressione dovrebbero per coerenza estendere la loro accusa di incostituzionalità all'intera disciplina in materia, la cosiddetta legge Reale-Mancino, che oggi è trasfusa nell'articolo 604-*bis* del codice penale, e dunque invocare sempre e comunque libertà di parola anche in materia razziale, etnica, nazionale o religiosa. Non lo fate perché qualche cognizione giurisprudenziale l'avete e sapete di avere contro tutta la giurisprudenza costituzionale, di Cassazione penale e quant'altro. Non è la propaganda di idee, ma l'istigazione a commettere atti discriminatori: tra i due concetti c'è, giuridicamente parlando, un abisso. Non deve trattarsi di semplici opinioni, ma di parole che, per portata istigativa, rischiano di tradursi o si sono tradotte in concreto in azioni discriminatorie, secondo uno stretto, diretto e consequenziale nesso di causalità. Ad essere punite non sono dunque le idee o le opinioni in sé, ma solo se in grado di trasformarsi in azione violenta e lesiva in concreto di un bene costituzionalmente protetto. Pertanto, occorre sempre «valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare altri a compiere un'azione violenta con riferimento al contesto specifico e alle modalità del fatto» (Corte di cassazione penale, sentenza I reati di istigazione a compiere atti discriminatori non si pongono dunque in contrasto con la libertà di espressione, perché «l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quanto meno intesa come comportamento generale, e realizza un *quid pluris*

Perdonatemi se ho citato tutta questa serie di sentenze e di citazioni giurisprudenziali, ma credo sia l'unico modo, l'unico argomento convincente per dimostrare quanto giuridicamente infondati siano, sotto questo profilo, sotto questo profilo, i timori espressi contro il disegno di legge Zan e come gli argomenti critici sollevati contro di esso, per loro valenza, dovrebbero indurre a rimettere in discussione l'intera legislazione penale contro i cosiddetti diritti contro l'eguaglianza ovviamente questa è una cosa impensabile. Non ci sono argomenti costituzionali giuridici fondati; solo una presa di posizione politica, legittima, ma completamente fuorviante e profondamente sbagliata. In altre parole, le ragioni della propaganda politica vorrebbero avere la meglio sulla ragionevolezza, sull'idea di eguaglianza e libertà costituzionalmente garantite. No, non si può proprio fare e non si può accettare. Per questo voteremo no alla questione

ribadiamo il nostro voto favorevole sulla questione sospensiva e ringraziamo sia la senatrice Malpezzi che il senatore Bressa perché ci hanno evidenziato tutta una serie di questioni molto complesse, sentenze della Corte costituzionale, della Corte POF e quant'altro, avvalorando la tesi che, essendo un tema molto complesso, il posto migliore per poterlo discutere è proprio la Commissione.

quella fu una proposta di riduzione del danno e non era volta a trovare una soluzione. Comunque ricordo a quest'Assemblea esattamente come votammo noi di Forza Italia la votazione finale sull'articolo 4 (ex articolo 3 alla Camera) fu una votazione di 242 a favore contro 171 contrari, quindi non proprio all'unanimità, Forza Italia, con il capogruppo dell'epoca Gelmini e il vice capogruppo vicario Occhiuto diedero indicazione di votare contro quell'articolo (è tutto nel resoconto dei lavori).

lo fecero proprio in virtù di quella riduzione del danno che aveva pensato l'onorevole Costa, sebbene noi continuiamo a dire che tale norma fosse comunque dannosa. Questo solo per ristabilire la verità. Aggiungo anche, se posso, che nella passata legislatura

di rivedere in Commissione al Senato e di migliorare questo testo. Se era giusto allora, perché non è giusto oggi, senatrice Cirinnà? Ce lo spieghi.

anche che il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa. Aggiunge inoltre, perché questo fa parte del *petitum* di almeno due proposte di questione sospensiva,

per cortesia, un attimo di silenzio, per rispetto del collega che vorrebbe intervenire. Lo dico immediatamente, per evitare ogni fraintendimento: l'intento della norma, signora Presidente e onorevoli colleghi, è decisamente giusto e va discusso senza ulteriori sospensioni, ma allo stesso tempo va difeso da ogni forma di intolleranza. Da un lato c'è una certa destra, che alla libertà di scegliere il proprio destino e alla libertà di amare preferisce sempre e comunque la legge del Vecchio Testamento, dall'altro però ci sono le intemperanze e le offese di chi vorrebbe addirittura che il Senato non discutesse alcunché. Ai primi voglio ricordare che la legge di Dio non è mai stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Quanto ai secondi, spesso minoranze emarginate e maltrattate, al fianco delle quali i socialisti hanno speso e lottato tutta una vita, si richiederebbe una dose di buon senso più alta, se necessaria a rendere la norma migliore. Sono state rivolte anche all'interno di quest'Aula - e a queste mi rifaccio - accuse monodirezionali, anche a chi vi parla. L'accusa principale è stata di voler rinviare *sine die* e di aver cambiato idea rispetto a un voto espresso alla Camera dei deputati. Io non ho cambiato nessuna idea e non voglio rinviare *sine die*, ma voglio esercitare il mio diritto di senatore a dire la mia, proprio perché chi ha guidato le battaglie civili in Italia, radicali e socialisti *in primis*,

non so se devo pagare il fio di essere stato decisivo nel voto della questione sospensiva, oppure il contrario. Mi ascolto volentieri, ma non avendo uno specchio, signor Presidente, gradirei perlomeno che lei ascoltasse, altrimenti mi posso sedere e consegnare il mio intervento alla Presidenza. È la prima norma di libertà all'interno di un'Assemblea.

vorrei ricordare che la vita delle battaglie civili dentro e fuori il Parlamento non è mai stata lineare.

Aggiungo che sulle unioni civili il percorso è stato altrettanto puntuto ed aspro: nel luglio 2014 è stato presentato un testo unificato, nel marzo 2015 un nuovo testo unificato, nell'ottobre 2015 un nuovo disegno di legge, nel febbraio 2016 un maxiemendamento con fiducia al Senato, l'11 maggio 2016 la Camera lo approva, dopo aver avviato una sua indagine conoscitiva. Stessa sorte per il divorzio breve, signor Presidente: approvato alla Camera nel maggio del 2014, al Senato un anno dopo nel 2015, di nuovo alla Camera in terza lettura ad aprile. Mai un percorso lineare. la prova di come - è quello che avviene anche all'interno dell'Aula - l'accusa equivalga spesso a condanna, tanto più quando viene amplificata dal tribunale dei *media.* appena proponi una modifica di civiltà - io ne ho una da proporre, quella che riguarda la libertà di opinione, resa incerta dall'articolo 4, nonostante l'ottima difesa fatta dal collega ed amico senatore Bressa - vieni paragonato alla destra tradizionalista, anche se hai speso tutta la tua vita in battaglie di civiltà, dal divorzio all'aborto fino alle unioni civili. I *social* raddoppiano le accuse, scatta la molla della vergogna, una presunzione di colpa di cui si avrà difficoltà per sempre a sbarazzarsi. Le modifiche che vengono proposte non appartengono soltanto alla destra, c'è anche una parte della sinistra di questo Emiciclo che chiede chiarezza sull'articolo 4.

come pecore rognose. Questa sarebbe la prova di una deriva illiberale, di una cultura che discrimina le opinioni differenti. Arrivo a chiedermi - e sarà questa la discussione dalla quale il dibattito sul disegno di legge Zan non potrà prescindere - se non si tratti di un ritorno a un certo ordine morale, proprio quell'ordine morale che venne spazzato via due secoli e mezzo fa dalla Rivoluzione francese e in quanto ordine morale non criticabile, benché una cosa sia criminalizzare l'istigazione alla discriminazione e altra cosa sia discriminare la propaganda. C'è di più: in un mondo segnato dal politicamente corretto, sono ancora più preoccupato per la libertà di espressione. Mi domando se sia davvero razzista chi non si inchina su un campo di gioco o se faccia una valutazione che prescinde dall'oggetto. Sia chiaro: nel disegno di legge Zan non c'è alcuna ingerenza negli affari della Chiesa e la lunga mano del Vaticano è stata una palese invasione di campo. Sia altrettanto chiaro che la norma Zan riempie un vuoto e se quel vuoto lo riempie, è un vuoto che va, dal punto di vista parlamentare, riempito. Voglio dare riconoscimento giuridico a minoranze che al momento sono state ignorate a lungo dal diritto e voglio sanzionare con severità gli atti di discriminazione e di violenza. però, cari colleghi e signor Presidente, è una società in cui la libertà di decidere e di esprimere la propria opinione sia garantita senza altri aggettivi. Non cito qui una marea di giuristi, di costituzionalisti ai quali spesso ci affidiamo in ogni lato di questo Emiciclo per supportare e sostenere le nostre opinioni. Ciò che non può accadere è che un'opinione personale - parlo dell'articolo 4 - venga sottoposta all'arbitrio decisionale di un giudice. Io non voglio che venga invertito un principio liberale, quello che seleziona solo le condotte vietate, mentre tutto il resto è considerato lecito. Il «purché» previsto nell'articolo 4 porta in questa direzione. Sarò ancora più chiaro e concludo: non voglio che si sostituisca una garanzia costituzionale, quella prevista dall'articolo 21 per la manifestazione del pensiero, con una garanzia da legge ordinaria. Abbiamo il tempo e il modo per chiarirlo e, se necessario, per sopprimerlo in Aula. La libertà non può essere sezionata a piacimento. Va bene per la legge Zan e non va bene per la libertà di opinione. *(Applausi)*. Lo dico soprattutto alla mia destra, ai compagni e agli amici del Partito Democratico, perché, se non riportiamo la libertà in questa fetta dell'emiciclo e la deleghiamo interamente a una destra retriva, veniamo meno a una funzione, che, cari amici e

l'onore, e in parte anche l'onere perché è una responsabilità importante, di iniziare il lungo elenco degli interventi di Fratelli d'Italia. Anzi, non è un elenco;

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Nel fondamento stesso del nostro ordinamento, dunque, non c'è spazio alcuno per tollerare discriminazioni o, peggio ancora, violenza, basate, tra l'altro, sul sesso dei cittadini o sulle loro condizioni personali. punisce ogni condotta penalmente rilevante che tragga origine da un pregiudizio discriminatorio. Vi è davvero un'esigenza concreta, reale e tangibile di legiferare in un campo già largamente disciplinato dalla legge anche penale e che trova richiamo nei principi della nostra Costituzione? Nella propaganda mediatica che accompagna il provvedimento si è usata la formula: "una legge contro l'odio". Ottima scelta comunicativa, ma sicuramente fuorviante, ancorché suggestiva: nessun reato consumato in Italia trova attenuanti o esimenti se motivati dall'odio. Invece, è esattamente vero il contrario. Il nostro ordinamento penale ha già tutti gli strumenti per sanzionare ogni atto tipizzato che sia commesso con intento discriminatorio, abietto e crudele. Incrementare le pene e le aggravanti già previste, come nello spirito del testo in esame, del resto, non rappresenta una risposta legislativa a un fenomeno particolarmente diffuso di delittuosità nei confronti di chi abbia sessualità cangianti, mutevoli o indefinite: tra il 2012 e il 2020 sono stati censiti in Italia 876 episodi di cosiddetta omofobia, come riporta il sito omofobia.org. 876 casi in otto anni rappresentano una media di 110 all'anno e di 9 al mese, a fronte degli oltre i 6.600 reati che vengono commessi e denunciati ogni giorno in Italia, con una media di circa 277 ogni ora. Da notare, peraltro, che di questi 876 episodi non tutti hanno rilevanza penale, in quanto spesso trattasi di accadimenti non denunciati oppure non necessariamente riconducibili a una forma di odio di genere; comunque, di certo non è sufficiente la mera querela per individuare in maniera definitiva la sussistenza di una colpevolezza aggravata dalla discriminazione. Dunque Dunque il testo si prefigge di normare ciò che è già normato, al fine di individuare aggravanti rispetto a ciò che è già aggravato, per incrementare la carica repressiva e punitiva di condotte già punite, solo per casi e situazioni di fatto numericamente limitati ed esigui, creando quindi una fattispecie peculiare che rende le vittime omosessuali di atti discriminatori più vittime delle altre. Tra gli elementi caratterizzanti del provvedimento in votazione è prevista la reclusione fino a diciotto mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi commette genericamente atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. È altresì previsto il carcere da sei mesi a quattro anni per chi istiga a commettere o commette violenza per gli stessi motivi o per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi. per qualsiasi reato commesso per tali finalità di discriminazione e di odio la pena viene aumentata fino alla metà. Francamente, non è comprensibile che il legislatore preveda tali aggravati strumenti sanzionatori in un ordinamento penale come il nostro, che riconosce e tutela tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, sanziona già ogni azione discriminatoria e punisce già severamente ogni condotta violenta, vieppiù se aggravata da motivi di odio, futili o crudeli. Con l'esclusione della richiamata identità di genere, peraltro, ogni altra previsione di discriminazione, odio e violenza è già largamente prevista dall'ordinamento; lascia molto perplessi quindi la genericità del provvedimento, che potrebbe prestarsi a difformi applicazioni da parte dell'interprete, sia nell'individuazione degli atti nella loro indeterminata accezione, sia rispetto al tema, i cui contorni sono ancora fluttuanti, della identità di genere. Ciò premesso, se è pur comprensibile un intervento, anche legislativo, finalizzato a rimuovere gli ostacoli che limitano l'eguaglianza dei cittadini, impedendo la libertà e il pieno sviluppo della persona umana, tale intervento deve appunto trovare la propria genesi nell'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione e non nella suggestione emotiva di alcuni accadimenti gravi, che pure sono accaduti e che trovano la nostra più ferma condanna. Compito del legislatore è una produzione normativa, a maggior ragione se penale, sempre ponderata e mai condizionata dalla spinta emozionale. Ancor più discutibile sarebbe una previsione penale e sanzionatoria distorta dall'ideologia, sorda ad ogni richiamo di saggezza pur di accontentare la velleità di una partigianeria culturale o di un gruppo di pressione. In linea di principio, comunque, è sempre un azzardo legislativo dividere e classificare le persone in categorie, proteggendone o tutelandone alcune più di altre, in quanto ciò finirebbe inevitabilmente per alimentare, implementare o acuire una disparità. L'attenzione verso soggetti deboli, fragili o maggiormente esposti, la cui situazione di pregiudizio o pericolo meritasse interventi normativi peculiari, non può, a sua volta, creare nuovi tipi di discriminazione o pregiudicare altri diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti. In tal senso, in verità, preoccupa molto il pericolo che il disegno di legge possa istituire limitazioni alla libertà di pensiero, una sorta di reato d'opinione la cui ricaduta appare oggettivamente antidemocratica e illiberale. L'articolo 4 del disegno di legge in discussione è sicuramente frutto di una posizione culturale inaccettabile, che, attraverso la repressione penale delle semplici idee, vuole istituire una polizia del pensiero. È oggettivamente impossibile, nel concreto, individuare con certezza preventiva quali espressioni del libero pensiero siano caratterizzate dalla idoneità a produrre un pericolo di compimento di atti discriminatori o violenti, specialmente se le maglie del dispositivo si allargassero a condotte eseguite astrattamente da parte di una pluralità indistinta di terzi. La libertà di parola, esimi colleghi, consiste proprio nel garantire a chiunque di poter esprimere idee non condivise, anche provocatorie o pungenti. Reprimere la libertà di parola significa soffocare il pensiero di chi non volesse adeguarsi alle posizioni dominanti. L'istituzione di censure e bavagli sfocia inevitabilmente nel regime autoritario. Non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo consentire che da quest'Aula venga istituita alcuna forma di limitazione della libertà di pensiero,

nessuno dovrà essere mai discriminato per i propri gusti o le proprie preferenze, laddove i comportamenti e le attitudini sessuali si svolgano in rapporti tra adulti consenzienti. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Tuttavia, non ci convincerete mai che da questo assioma che, lo ripeto, ci trova assolutamente favorevoli, possa scaturire un modello di società repressiva contro le libere opinioni.

Preliminarmente, voglio dire che ho sbagliato a fotografare il collega Faraone, benché questa sia ormai una pratica molto diffusa. Ammetto l'errore, ma resta il mio giudizio politico. Ognuno è libero di applaudire, ma ognuno è libero di dare significato politico alle singole azioni. signor Presidente, colleghi, non sarà facile né troppo breve questo mio intervento, il primo del Gruppo del Partito Democratico, Gruppo titolare e firmatario di questa legge.

Si occupa di dare piena attuazione all'articolo 3 della Costituzione, una norma fondamentale sulla quale non dovrebbero esserci differenze tra di noi. Eppure, ci sono e ci sono state molte differenze, a cominciare dalla Commissione giustizia del Senato, una Commissione che ha ostacolato, attraverso l'operato del suo Presidente, il lavoro su questo testo fin dall'inizio, addirittura rimodulando 170 audizioni, ripercorrendo anche quelle fatte alla Camera.

è una cosa inaudita. E quando si è sbloccato l'incardinamento? Si è sbloccato quando il dibattito pubblico, quando il dibattito sui *social*, quando quegli *influencer*, che tanti blandiscono ma che, secondo me, tanti temono, hanno alzato il tiro sul perché il testo non venisse incardinato. Penso anche alla grande mobilitazione del mondo LGBT e del mondo femminista, culminato in un grande appello di 114 associazioni che ci chiedono che questo testo sia approvato senza modifiche. 114 sigle ci chiedono che questo testo sia approvato senza modifiche. Il movimento LGBT italiano, in modo praticamente unitario, dice: «Meglio nessuna legge che una cattiva legge». che cosa il testo Zan interviene, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. Esso punisce i reati d'odio, estendendo fattispecie già previste dalle nostre leggi, in particolare dalla legge Mancino. Non è vero che si introducono nuovi reati; si estendono fattispecie di reato già esistenti, che sono il compimento di atti discriminatori e violenti e l'istigazione a commetterli. Non viene esteso il reato di propaganda delle idee; ripeto, non viene esteso il reato di propaganda delle idee, che resta limitato alle idee fondate sull'odio razziale e sull'odio etnico. Questi reati, già previsti, vengono estesi per proteggere alcune fondamentali dimensioni della personalità (sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità) e, per le stesse ragioni, viene estesa la circostanza aggravante speciale della legge Mancino. Cari colleghi di Forza Italia, non ci accontentiamo dell'aggravante semplice dell'articolo 61; abbiamo bisogno di tutele più forti per queste soggettività.

chi lo dice forse vuole continuare a essere libero di spargere odio e alimentare violenza. No, non è così. Il disegno di legge Zan non si occupa assolutamente di regolare la circolazione delle idee nello spazio pubblico di questo Paese; si occupa soltanto di proteggere la dignità delle persone, punendo solo le condotte idonee a determinare un concreto pericolo di violenza o di discriminazione. di legge Zan mette in campo per applicare l'articolo 3 della Costituzione è fare cultura. Quante volte abbiamo sentito dire in quest'Aula che la violenza non si può fermare soltanto

celebrata in luoghi pubblici e anche nelle scuole. Voi dite che lo fa ideologizzando i bambini, una *fake news* meschina e degradante. Ai giovani, come ha spiegato perfettamente la presidente Malpezzi - si cercherà solo di far capire, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, per cui le scuole potranno e non dovranno - che le differenze esistono e che devono essere rispettate e questo non lo chiede Monica Cirinnà, strega, eretica e pericolosa; lo chiede la Costituzione che promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, unico modo per contrastare il bullismo. legge Zan si occupa di questo e di nient'altro. Ogni nuova *fake news* è una coltellata alla dignità delle persone LGBT: troppe volte lo abbiamo visto. Con il mio personale e grandissimo dolore, presidente La Russa, abbiamo sentito nelle audizioni un ex magistrato equiparare l'omosessualità alla pedofilia: continue coltellate alle persone più fragili. Pochi passaggi per ricordare l'*iter* parlamentare lunghissimo di questo provvedimento. Tra l'altro, grazie al collega Zan, che ha accolto un suggerimento, abbiamo tenuto per oltre un anno una bicamerale informale tra componenti delle Commissioni giustizia del Senato e della

ha molto lavorato. Penso alla grandissima generosità della presidente Laura Boldrini, che ha fatto confluire il suo testo contro la misoginia all'interno

ha introdotto, chi voleva ha ottenuto. Oggi però, proprio sui punti su cui abbiamo lavorato a lungo alla Camera, qualcuno chiede di nuovo discussione. Su cosa dobbiamo ancora discutere oggi? Abbiamo mediato sull'identità di genere; abbiamo mediato sulle scuole; abbiamo mediato sulla libertà di manifestazione del pensiero. Quali altre mediazioni sono necessarie? Quali sarebbero le ragioni di merito per cui, avendo già votato questo testo alla Camera, cambiare idea adesso? A me pare chiaro che sulla pelle delle persone LGBT si sta giocando un'altra partita; sulla pelle del movimento; sulla pelle delle persone diversamente abili; sulle migliaia di donne colpite da misoginia. Questo gioco politico tattico non fa bene alla politica Voglio chiudere il mio intervento portando in quest'Alula la voce delle persone trans, protagoniste ignorate di questo dibattito. Sono mesi che discutiamo di identità di genere, ma lo stiamo stiamo facendo, colleghe e colleghi, senza ascoltare la voce delle persone interessate, che chiedono protezione allo Stato per il modo in cui vivono la propria identità di genere, che troppo spesso le espone alla discriminazione e alla violenza. Ci stiamo occupando Ci stiamo occupando di un testo giuridico, colleghi, non antropologico, sociologico o di filosofia. Stiamo solo provando a dare protezione a persone discriminate dalla violenza. Per questo voglio citare le parole di Porpora Marcasciano, storica attivista trans, una persona che - vi piaccia o no - ha fatto la storia di questo Paese, tracciando cammini nuovi per la libertà di tutti

«Mi chiamo Porpora Marcasciano, sono presidente del Movimento italiano dell'identità trans (MIT), attivista militante del Movimento LGBT+ dagli anni Settanta. La mia voce è la stessa di 400.000 persone trans (la stima è dell'Istituto superiore di sanità, ferma al 2019) e ora più che mai vi chiedo di non bloccare il disegno di legge Zan: esso arginerebbe soprusi e violenze che quotidianamente siamo costretti a subire. Prima di pronunciarvi, vi chiedo di comprendere, o quantomeno di approfondire, il significato che ha per noi la frase "identità di genere". Nessuno ci ha convocato, nessuno ci ha ascoltato; e i nostri vissuti non vi sono arrivati. Lo avremmo gradito, perché state legiferando sulle nostre vite. Pensate che l'Italia, secondo le statistiche più recenti, è al primo posto in Europa per numero di vittime di transfobia. I trans italiani chiedono ai parlamentari di adeguarsi ai tempi e guardarsi intorno, soprattutto ai Paesi cosiddetti avanzati e civili, le democrazie di cui tanto ci sciacquiamo la bocca. Dare a noi non significa togliere ad altri, significa dare a noi e a tutte e tutti una società più bella e più giusta». Ecco le parole di Porpora Marcasciano; ecco la spiegazione,

chi chiede mediazioni ora non è più credibile. Siamo ormai fuori tempo massimo. Chi vuole giocare al gioco della torre? Chi vogliamo buttare giù? Le persone trans o in transizione, escludendo la definizione di identità di genere e lasciandole senza protezione? Oppure vogliamo buttare dalla torre l'articolo 4, lasciando i peggiori odiatori - fuori e dentro i *social* - liberi di calpestare la dignità delle persone fragili? O infine vogliamo buttare dalla torre l'educazione, la cultura, la possibilità che nelle scuole si possa scegliere cosa insegnare ai nostri ragazzi? No, colleghi, noi non giochiamo al gioco della torre, non lasciamo indietro nessuno. Vogliamo che questa legge sia approvata così com'è, per proteggere tutte le persone dalla violenza. Senatrice Cirinnà, come ha potuto rilevare, la passione del suo intervento - al di là dell'adesione o meno - ha consentito che le venisse riservato un tempo maggiore di quello che è stato riservato

Di questo realmente si tratta, dietro la maschera del dare una protezione a chi oggi, di fatto, già ce l'ha. La prova della correttezza del mio convincimento sta proprio in quell'infelice articolo 4, che molto ha colpito e che letteralmente recita: «(*Pluralismo delle idee e libertà delle scelte*) 1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte». Sono fatte salve: e da chi? Da un disegno di legge? È fatta salva la nostra libertà di espressione e di opinione? Che sia stato abrogato l'articolo 21 della Costituzione non ce ne siamo accorti. Non avevamo certo bisogno di un disegno di legge per vederci riconosciute le nostre sacrosante libertà. Lo ha già fatto per noi la legge delle leggi, che è la nostra Carta costituzionale. E, come se non bastasse, è inutile una simile clausola di salvezza, che, sempre nel corpo dello stesso articolo 4, è seguita da una pericolosissima previsione, e cioè che libertà sono fatte salve purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Mi domando e vi domando: chi decide circa l'idoneità a determinare il concreto pericolo? È chiaro che a decidere sarà la magistratura. Avete una vaga idea di quanta discrezionalità stiamo decidendo di consegnare nelle mani dei giudici? Credo che non sia giusto. A fronte di cosa, poi? Perché dovremmo pagare questo prezzo così alto? Forse perché Zan e i suoi alfieri che vanno in televisione ci vengono a raccontare dell'urgenza della repressione di questo pseudo-pericolo dell'omofobia? Ci incalzano e ci dicono che dobbiamo fare in fretta, perché è una questione di vitale importanza.

perché dovremmo pagare questo prezzo così alto? Forse perché Zan e i suoi alfieri vengono a raccontarci che è un provvedimento di vitale importanza, per cui ci incalzano e ci dicono che dobbiamo fare in fretta? E, alla luce di questa presunta vitale importanza, E, alla luce di questa presunta vitale importanza, ci propinano di fatto un disegno di legge fatto male, scomposto e con effetti collaterali, sbandierando ai quattro venti statistiche assai dubbie e molto poco ufficiali, così com'è stato anche rilevato da colleghi che mi hanno preceduto. Dobbiamo avere chiaro che, ove passasse mai una siffatta norma, sarebbe in pericolo la possibilità che ognuno abbia la propria idea sugli omosessuali e sui transessuali, sulla transessualità. Con il tipo di giustizia che c'è in Italia, si correrebbe financo il rischio che un'associazione possa querelare per incitazione all'odio laddove qualcuno si avventurasse ad esprimere la più banale delle affermazioni, come quella per cui il matrimonio è soltanto quello tra uomo e donna. Si rischierebbe persino per tale via di portare in tribunale una marea di opinioni che non sono assolutamente istigazioni all'odio. È inutile: il disegno di legge Zan non serve; abbiamo già leggi che vietano l'aggressione fisica e bisognerebbe soltanto farle applicare, come avviene per tante altre, che ci sono e non vengono applicate. Credo che non abbiamo bisogno di ulteriori distinzioni e discriminazioni tra esseri umani; abbiamo bisogno di più cultura sociale e di più senso civico: non si picchia un essere umano a prescindere e non perché è *gay*, disabile o la sua pelle ha un colore diverso dalla nostra. Non è più grave, se si picchia una lesbica piuttosto che una donna. È grave picchiare e l'aggravante dei futili motivi è già presente nella nostra normativa. È possibile che convenga a molti avere queste differenze, a quanti trovano in questo modo una ghettizzazione proficua, forse anche anche economicamente. Evidenzio che in molti Paesi, nel Nord Europa, non ci sono più le strade e i locali *gay* o i rioni cosiddetti arcobaleno. Vorrei vivere in un Paese dove gli uomini e le donne sono uguali e i locali sono per tutti - *gay*, etero o lesbo - senza ghettizzazioni Non sarà con il disegno di legge Zan che educheremo la nostra società all'integrazione, all'accettazione e all'accoglienza del prossimo. Per far ciò è necessaria una rivoluzione copernicana, che coinvolga le principali agenzie educative e sia condivisa, e pacifica, che parta dal rispetto del riconoscimento dell'altro, alfabetizzando emotivamente i nostri giovani, affinché compiano un salto evolutivo da istinto ad emozione e da emozione a sentimento. saremo tutti uguali, non avremo più bisogno della *gay street* accanto al Colosseo a Roma, ma avremo città aperte in egual modo, senza veramente discriminare nessuno. Desidero condividere con voi altre preoccupazioni e preoccupanti osservazioni, che ho maturato sul disegno di legge in discussione. Penso in particolare al tema del o autopercezione di genere, che ha già procurato moltissimi problemi dov'è in vigore. Gli esempi di questo impatto di genere sulle donne sono innumerevoli. Si pensi a quanto è successo in California dove, in forza della nuova legge sul *self-id*, quasi 300 detenuti maschi che si autopercepiscono donne hanno chiesto di entrare nelle carceri femminili, terrorizzando le detenute. In Canada, dove questa cosa è già successa, si sono verificate violenze sessuali o addirittura gravidanze e casi di malattie sessualmente trasmesse. Si pensi inoltre ai corpi maschili coinvolti in competizioni competizioni sportive femminili. Non se ne parla sui giornali, eppure alle prossime Olimpiadi la questione potrebbe deflagrare. Sempre in base al *self-id*, vari uomini occupano cariche politiche e, in generale, posti di lavoro che in base alle quote rosa dovrebbero essere riservati alle donne. Anche in questi casi, cresce la percentuale di aggressioni sessuali commesse da uomini che si identificano come donne. Questo accade negli altri Paesi da quanto detto, non mi pare che ci si trovi al cospetto di una buona pratica che merita di essere replicata in altri ordinamenti, anzi, direi proprio che forse è il caso di fare tesoro di tali inadeguatezze e disfunzionalità per rimanere ben lontani da tali cambiamenti, che non migliorano il sistema, ma lo abbrutiscono. Lasciatemi infine spendere le ultime osservazioni sull'articolo 7, che in un colpo solo mette a rischio la libertà di insegnamento, il primato educativo dei genitori e l'istruzione dei minori. di contrastare discriminazioni per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, in realtà il disegno di legge Zan dimostra che lo scopo è di favorire l'ideologia *gender*, l'ideologia *gender*, che nega la dimensione sessuata dell'essere umano e considera la naturale differenza fra uomo e donna una mera costruzione sociale. il disegno di legge parla di identità di genere, espressione che indica il senso di appartenenza di una persona a un genere con il quale essa si identifica a seconda di come si percepisce in un dato momento (fluidità del genere). Ebbene, la primazia della scelta educativa genitoriale non solo è prevista all'articolo 30 della nostra Carta costituzionale, ma è finanche sancita a

È chiaro che tali convinzioni filosofiche, religiose e pedagogiche devono essere lecite e degne di tutela secondo le istituzioni del Paese membro. Se, come genitore, non volessi che a mio figlio venisse insegnata la cultura *gender,* educandolo piuttosto al rispetto di tutte le diversità, lasciando fuori dal momento educativo tematiche

di genere tendano a emergere nei gruppi di ragazzini per imitazione: già abbiamo l'anoressia per imitazione, mi sembra il caso di riflettere. Ho ascoltato con molta attenzione il presidente Ostellari, che ci ha messo a conoscenza dell'*iter* che il provvedimento ha avuto

a un muro contro muro, onestamente non me lo spiego. La Conferenza dei capigruppo ha deciso che si potranno presentare gli emendamenti e mi auguro che si creino le condizioni per accogliere le ragioni di tutti, che si trovi il modo per sedersi intorno a un tavolo e che con il confronto si possa accogliere e non respingere; se si arrivasse a votare all'unanimità il disegno di legge in esame, modificandolo, sarebbe un bel segnale. Spero davvero che la conclusione di questa vicenda possa eliminare inutili contrapposizioni ideologiche. Mi rivolgo in modo particolare all'onorevole Letta, che è erede della tradizione cattolica democratica di Aldo Moro e allievo di Nino Andreatta; spero non continui a irrigidirsi, mandando a gambe all'aria una cultura e una storia fatte di distinzioni, sì, ma anche di rispetto. La fatica della democrazia richiede confronto e vocazione La fatica della democrazia richiede confronto e vocazione all'intesa, soprattutto quando ci sono in campo principi e valori diversi. Su questi aspetti, per così dire, sovrapolitici occorre sempre una mediazione alta, che non è compromesso al ribasso. banditi sovranismi e dogmatismi, mentre occorre recuperare quel saggio realismo moroteo del possibile, che si fa carico dei punti di vista degli altri per approdare a una confluenza tra distinti. Nel caso si decida, sbagliando, di respinge gli emendamenti, creando un'illogica situazione fuori dalla logica morotea a cui molti di noi ancora s'ispirano e a cui tanti ancora fanno riferimento, mi vedrò costretta a votare contro. *(Applausi)*. Governo, onorevoli colleghi, nei miei interventi in quest'Aula sono sempre stato molto moderato e possibilista, ma oggi su questo argomento intendo dire tutto quello che penso. Spero di poter invecchiare, finita questa esperienza, e passeggiare nelle strade della mia provincia senza essere insultato da coloro che non sono d'accordo con il disegno di legge in discussione. Mi spiego meglio: tutte le persone che ho incontrato in queste ultime settimane e non frequento cattive compagnie, ma gente normale (cattolici impegnati, elettori di destra e di sinistra, gente che lavora) - mi hanno espresso la loro contrarietà ai concetti del disegno Tutti. Forse non riesco a frequentare proprio quegli altri che la pensano secondo quanto dichiarato poc'anzi (quelle 135 associazioni). di legge Zan non è emendabile, perché, se togliamo l'identità di genere dall'articolo 1, la discrezionalità del giudice troppo elevata e l'educazione scolastica, non ci resta più niente;

Ci sono nuovi teorici alla moda, come Fedez, e la *lobby* LGBT, che è molto potente, soprattutto in televisione e in parte della cultura, e che ha partorito un testo che va oltre le necessità e i bisogni da tutelare. Ne spiego i motivi. Si legifera su temi che sono prepolitici: la società esisteva prima della nascita dello Stato. La famiglia esisteva prima e si regolamentava nei suoi rapporti: penso al diritto naturale o alla stessa psicologia, conscia o inconscia. La crescita dei bambini, la nostra crescita, è stata discreta e graduale nell'ambito della famiglia, soprattutto su certi valori. Pensare che lo Stato debba educare su tutto è un concetto comunista, che vige in Corea del Nord e forse in pochi altri Stati.

C'è semmai una visione che è attinente alle concezioni religiose; tra l'altro, anche i musulmani o parte di loro (è una struttura molto complessa quella musulmana) sono contrari a questa legge. Secondo la religione cattolica - nello spirito di Benedetto Croce, non possiamo non dirci cristiani - c'è una dottrina tratta dalle Lettere di san Paolo, o il Magistero di Wojtyla e Ratzinger (cito quelli che, secondo me, sono nella completa e perfetta ortodossia), secondo cui i principi non negoziabili della Chiesa ci sono.

- anche su questioni che apparivano non troppo significanti per apparire moderni, conformi ed essere osannati dai laici e soprattutto dai laicisti, ha portato la Chiesa a può esprimersi soltanto al riguardo di quello è scritto nel Concordato, che è importante, ma non è la sostanza, bensì la forma. Oggi la Chiesa si è ridotta a essere fondata sull'ambientalismo e sull'accoglienza, dimenticando la dimensione verticale ed escatologica. Ciò è molto grave e speriamo che ci sia una scuola, tipo quella dei monaci del Medioevo di Cluny, che faccia riprendere forza e vigore alla Chiesa, tanto quanto merita. Anche tanti *gay* che conosco, che vivono singolarmente o in coppia, sono contrari a questa legge. Vivono con dignità e rispetto

delle teorie *gender* e di ciò che comportano nell'educazione e nelle trasformazioni, anche radicali, dei bambini sono quasi contro natura, secondo la mia concezione. La discrezione del giudice, come già detto, nelle opinioni, *ex* articolo 4, è troppo ampia e sarà pericolosa. si possano mettere al posto del proletariato, che era al centro delle attenzioni dei partiti di sinistra, i *gay* e i *gay* e questi argomenti? Pensate che chi rappresenta queste tendenze sia più intelligente? Voi pensate - o una parte di quelli che sono a favore che il Governo sia soltanto di certi partiti e non degli altri, che sono accolti, ma solo come parenti poveri, perché hanno una macchia dalla loro nascita? Non è così. Che società vogliamo?

Se fossimo tutti così, non ci sarebbe più natalità. E allora perché la difendiamo? Una società simile, secondo la vostra concezione, è immersa in problematiche socioassistenziali, create e mantenute all'infinito, al fine di favorire le associazioni che percepiscono i contributi pubblici (vedi l'immigrazione e i nuovi centri previsti dall'articolo 8 del disegno di legge Pensate che ci sia una società che si diverte. E come vive? Vive secondo i concetti tradizionali, quelli dei nostri Paesi e delle nostre comunità. Come si diverte? Si diverte in modo normale e ci sono tante cose belle e interessanti, se fatte bene. È una società che produce, cresce e paga il debito, quando è così confusa? Per mio conto, la legge Zan è la prosecuzione di un concetto e di un disegno nichilista della società; poi ci sarà l'eutanasia (c'è già un disegno di legge che circola). Ci sono gli stessi sintomi, a mio avviso, della caduta dell'Impero romano. Con tutte le forze, pertanto, credo ci siano anche nello schieramento favorevole persone che sono in crisi di coscienza e che hanno una storia come la mia e come tanti di quelli che votano no. Voterò no in tutti i modi, così come farà Forza Italia, lasciando tuttavia libertà di coscienza, come ha sempre predicato Berlusconi. Vi invito a meditare su quello che si va eventualmente a decidere con maggioranze risicate: è una questione che va approfondita e, semmai, approvata a maggioranze larghe, come si sta facendo su altri argomenti, tutti importantissimi, soprattutto in questo momento momento di crisi e di trasformazione della società. Approfitto della possibilità di avere ancora mezzo minuto per ripetere che sono fermamente contrario anche a una modifica. Questa legge non può passare.

questo non è un disegno di legge: questo è un disegno di nuova umanità. Si vuole utilizzare una battaglia giusta e condividibile, quella contro ogni forma di aggressione ingiustificata, facendola diventare un grimaldello per trasformare le basi stesse della nostra società. Vediamo se riesco a dimostrarlo nei minuti che mi sono stati concessi. È un disegno di uomo che è denunciato già dall'articolo 1, dove si vanno a sostituire parole naturali come «sesso», previste dalla nostra Costituzione e semplicemente dalla naturalità dell'essere umano, con «genere», «orientamento sessuale» e «identità di genere». Cos'è l'identità di genere? Credo che molti in quest'Aula ignorino cosa sia davvero l'identità di genere. Questa, attualmente codificata per esempio sul sito Facebook, ammonta a 58 identità differenti che, oltre al maschile e al femminile, anche *gay*, lesbica, bisessuale, transessuale, *transgender*, *cisgender*, *queer*, pansessuale, intersessuale, genere non binario, *genderqueer*, androgino, asessuale, *agenderflux*, demisessuale, *grey asexual*, aromantico. E potrei continuare per ore. Siamo davvero convinti che presentare ai nostri figli l'alternativa tra queste identità di genere sia un buon modo per crescerli liberi, sereni ed equilibrati? Credo che che offrire tutte queste identità di genere serva in realtà a togliere l'identità ai nostri ragazzi, ai nostri figli. Vorrei leggere le parole di Keira Bell, una ragazza inglese che ha fatto una transizione di genere quando aveva sedici anni. È stata convinta nella sua scuola a fare una transizione e quindi si è fatta amputare il seno e si è fatta trasformare i genitali, dopo un lungo periodo di trattamento con con bloccanti della pubertà. Le sue parole, dopo aver vinto la causa contro la clinica Tavistock and Portman di Londra: «Non si possono prendere decisioni simili a sedici anni e così in fretta. I ragazzi a quell'età devono essere ascoltati e non immediatamente assecondati. Io ne ho pagato le conseguenze, con danni gravi fisici. Ma così non va bene, servono cambiamenti seri». Questo sta accadendo non in ignoti Paesi del terzo mondo, ma nella civilissima Londra, nella civilissima Gran Bretagna, dove anni fa è stata approvata una legge, l'Equality Act, che è molto simile al disegno di legge Zan. Grazie all'Equality Act, ogni forma di resistenza da parte dei medici, del personale ospedaliero, degli insegnanti e degli stessi genitori alla transizione di genere dei minorenni è stata etichettata come omofobia. Siccome non mi credete, vi invito a leggere alcuni libri. Sono in lingua inglese, perché ovviamente non vengono tradotti in italiano. «Christians in the firing line», per esempio, scritto dal dottor Richard Scott, racconta come, sempre nella civilissima Gran Bretagna, un magistrato abbia perso il lavoro e sia stato licenziato semplicemente per aver scritto in una sentenza che i bambini, in caso di adozione, hanno il diritto di essere adottati da una coppia con mamma e papà e non da una coppia di persone dello stesso sesso. È stato licenziato e il suo nome è Andrew McClintock. Non solo: c'è un altro caso - potrei andare avanti per ore a leggerveli - di un medico pediatra di comunità che ha perso la causa contro il servizio sanitario inglese ed è stato licenziato per aver dimostrato scientificamente che i bambini crescono meglio in un contesto in cui la genitorialità è costituita da mamma e papà.

che è un interessantissimo testo in inglese sulle ideologie che vengono utilizzate per indottrinare i ragazzini, fin dall'età più piccola, in cui si va sostanzialmente a insegnare che qualunque tipo di sensazione qualunque tipo di sensazione del bambino dev'essere immediatamente assecondata e seguita. Vorrei raccontare in quest'Aula la storia di un papà canadese, che si chiama Robert Hoogland. Avete tutti Google e potete cercare il suo nome: Robert Hoogland non si è rassegnato al fatto che la sua bambina, alla scuola superiore, all'età di dodici anni - quelle che da noi sono le medie, in Canada sono già superiori - fosse stata convinta nella sua scuola a cominciare la transizione di genere. Egli si è sempre rifiutato di assecondarla, perché riteneva che fosse sbagliato. Il giudice, non più tardi di due mesi fa, lo ha condannato a sei mesi di reclusione e a 30.000 dollari di multa semplicemente per aver usato verso sua figlia il pronome femminile *she* e aver continuato a chiamarla con il suo nome da bambina. Quella era la sua bambina. Queste non sono invenzioni, ma storie di Paesi che hanno seguito prima di noi questa strada e ora stanno tornando indietro. Tavistock and Portman di Londra ora è sotto attacco giudiziario e la metà dei medici di quella che era una delle cattedrali mondiali del *gender* si è dimessa.

inoltre un problema enorme dal punto di vista della libertà di parola. Ho già raccontato in Commissione - e vorrei farlo anche in quest'Aula - la storia di un pastore protestante, di nome

discriminata e ha fatto appello all'Equality Act, chiamando la polizia, che è intervenuta, lo ha arrestato e ammanettato, trascinandolo via in mezzo alla folla. Vi prego di guardare su Internet il video dell'arresto di John Sherwood, che è stato trattenuto per ventiquattr'ore alla stazione della polizia e ora è sotto processo per omofobia. Pensate forse che queste cose non accadranno? È chiaro che in questo momento tutti vi raccontano che la libertà non è assolutamente in pericolo e, anzi, potrete continuare a dire di essere contro l'utero in affitto.

perché la propaganda è un discorso e i vari Fedez di turno sono un altro, ma qui dentro le cose dovremmo avere il coraggio di vederle non solo con gli occhi delle ideologie o con gli occhiali del partito politico di appartenenza, ma con la testa di chi sa vedere quali sono le conseguenze che in altri Paesi hanno generato ingiustizie

questa frase sarà discriminatoria, perché ci sono i cosiddetti papà cavalluccio marino, che in realtà sono donne, che però hanno fatto la transizione, bombardandosi di ormoni, e quindi hanno la barba, i peli e tutto quello che serve per essere uomini, tranne i genitali, che hanno mantenuto femminili; a quel punto, possono restare gravide, ma vogliono essere chiamate "papà" e chiamarle mamme o donne diventerà automaticamente discriminazione. Andate a vedere che cos'è successo alla madrina di Harry Potter, l'autrice inglese Rowling, che si è permessa di scrivere su Internet che la parola «donna» non può essere sostituita dalla definizione «individuo che mestrua», perché quell'espressione è discriminatoria verso la donna. Ha osato dire queste parole. Ebbene, è stata bombardata e massacrata sui *social media*, perché si è detto che non rispetta gli uomini che mestruano. Siamo a questo? Siamo al punto di non sapere più distinguere il maschile dal femminile? Guardate che poi queste non saranno bizzarre teorie che il senatore Pillon agita in Aula, spaventando la folla degli astanti: diventeranno sanzioni penali e sono pronto a giurare in quest'Aula che un giudice in in Italia - ma saranno più di uno - condannerà qualcuno, perché ha osato dire che le donne hanno il ciclo mensile e i maschi no. Sarà considerata grave discriminazione. Ancora, avete letto gli articoli 5 e 6 di questo Avete letto le pene accessorie folli per chiunque osi discriminare o istigare alla discriminazione sulla base dell'autonomia di pensiero di chi si sente uomo, anche se è donna? Ebbene, le pene accessorie, oltre alla galera, sono anche

politica e ovviamente quello alla patente di caccia, ma addirittura la propria dignità, perché sarà costretto a fare lavori socialmente utili presso le associazioni LGBT, per la pena del contrappasso. Questo prevedono gli articoli 5 e 6. Avete letto

come faranno i genitori? O faranno la scuola a casa, cioè la scuola parentale, o dovranno tenere i figli ignoranti. *(Applausi)*. Cara senatrice Malpezzi, siamo capaci anche noi di leggere, ci creda sulla parola,

della Regione Lazio, che sono state precipitosamente ritirate, nelle quali c'era scritto che è buona prassi assecondare i ragazzi nella transizione, ovviamente fin dalla più tenera età, e addirittura garantire la carriera *alias*.

e deve andare nel bagno delle donne. Questa vi sembra una cosa normale? Vi sembra una cosa giusta? *(Applausi. Commenti)*. Benissimo. Siccome giustamente voi ammettete che questa è una cosa giusta

tutto qui: «Fiabe d'altro genere». Vi invito a leggere questo libricino, che sarà sicuramente utilizzato, insieme a molti altri che non ho portato in Aula. E visto che pensate che sia assolutamente giusto tutto ciò, vi invito a leggere le parole dei genitori tedeschi che sono stati arrestati per aver rifiutato di portare i loro figli a scuola perché quel giorno c'era la lezione di

dov'è la libertà di scelta dei genitori? Dov'è la libertà di educazione prevista dall'articolo 30 della Costituzione? *(Applausi)*. Come sempre, ci sono due bei pesi e due belle misure.

sono stati così sfortunati da avere perso la loro mamma e il loro papà. Il meglio significa costruire le condizioni perché trovino una coppia, mamma e papà, che il più possibile assomigli alla coppia che è stata tolta loro dalla natura, dal caso o da una disgrazia. Noi, invece, andiamo a sostituire e, quindi, aumentiamo il danno e usiamo persone già di per sé sfortunate per fare esperimenti sociali; e poi scopriamo che questi esperimenti sociali falliscono, ma non si può dire

la mamma è femmina, che genitore uno e genitore due non è giustizia sociale, non è equità, non è rispetto. *(Applausi)*. Prima dobbiamo rispettare i bambini; poi rispettiamo gli adulti.

una nuova umanità in cui tutto sarà famiglia perché, a quel punto, due uomini saranno famiglia e due donne saranno famiglia. A quel punto, perché non tre o quattro? Sarebbe discriminatorio e, quindi, tutto sarà famiglia e niente più sarà famiglia. Non esiste una società che sia sopravvissuta alla distruzione della famiglia. Non esiste. Non so cosa accadrà in questa Aula. I numeri di oggi fanno molto ben sperare che tanti colleghi abbiano compreso che c'è una preoccupazione che va giustamente assecondata, ma che, d'altro canto, però, non si può ignorare una pericolosa deriva ideologica. Se tutto diventa famiglia e, quindi, niente più è famiglia, la società diventa un coacervo di individui non più di persone. Arrivo alla conclusione del mio ragionamento non senza avervi segnalato un ultimo libro. tratta di un *report* che è stato presentato al Senato due settimane fa sulle violazioni delle libertà fondamentali causate dalle leggi sulla omotransfobia. Sono tutti casi estremamente concreti, documentati, in cui si evince come il pericolo che leggi simili al disegno di legge Zan si trasformino in un una sorta di *boomerang* per la libertà civile, per la libertà di educazione, per la libertà di pensiero, per la libertà di parola, per la libertà di culto assolutamente concreto. C'è una simpatica storia, che ho pubblicato anche sul mio canale, che racconta di un signore transessuale, un maschio, che ha chiesto di entrare in un convento di clarisse in Belgio. Sembra una barzelletta, invece è una storia vera. Questo signore si è sentito discriminato d'altronde l'unico motivo per cui sono state rifiutate la sua iscrizione e la sua adesione a questo convento di clarisse è che era un maschio; quindi oggettivamente è stato discriminato in base al suo sesso. C'è anche un altro caso di una signora alla quale è stato negato l'ingresso in un seminario cattolico e l'unica ragione per cui è stata esclusa è che era femmina e non c'è un'altra ragione; quindi, è vero, è stata discriminata in base alla sua identità sessuale. Ma siamo convinti che sia tutto uguale, sia tutto identico, sia tutto allo stesso livello, sia tutto possibile? Siamo convinti che qualunque tipo di scelta, sulla base di una visione antropologica fondata sulla naturalità della differenza maschile e femminile o - volendo fare il Pillon a tutti i costi - una visione fondata sulla propria fede religiosa non abbia più libertà di essere definita, raccontata, vissuta e non abbia più la libertà di diventare anche una tradizione, un modo di vivere la società? Io sono convinto che questo sia il più grande errore che noi possiamo fare. La società non si è costruita ieri e non è che sono arrivati i teorici del *gender* a scoprire che il maschile e il femminile sono la causa di tutti i disastri, di tutte le ingiustizie del mondo e che quindi vanno "spianati"

non dobbiamo darci come limite quello di una legge a tutti i costi. Penso che abbiamo una possibilità concreta, che è quella di affrontare il fenomeno,

chiunque minaccia, chiunque provoca lesioni personali, chiunque attenta alla vita di qualcun altro, chiunque ingiustamente licenzia, chiunque ingiustamente esclude:

Qui c'è un'Assemblea che è divisa perché si è voluta inserire una ideologia inaccettabile in un disegno di legge che aveva un altro scopo. Tutti noi abbiamo esultato per l'Italia che ha vinto la finale degli Europei. È stato interessante vedere qual è stata la prima reazione dei nostri beniamini, dei giocatori. Non hanno telefonato al genitore 1 o al genitore 2. Hanno chiamato la mamma! Hanno chiamato la mamma e le hanno detto: ciao mamma, guarda quanto sono stato bravo. Ho vinto. Noi italiani abbiamo degli anticorpi preziosi contro queste ideologie che ci vengono da una visione dell'uomo maturata nei *college* universitari del Nord America. Perché queste ideologie hanno un nome e un cognome: si chiamano Judith Butler, si chiamano Donna Haraway, di filosofi e antropologi convinti che solo dal superamento del binarismo sessuale maschile e femminile avremo una società più giusta. Non è così! Andate, vi prego, a vedere la società svedese e le società del Nord Europa, dove tutto questo è già realtà. Ve lo ripeto. L'ho già detto e lo dico ancora una volta. Abbiamo questa possibilità. Siamo un passo indietro e ancora non siamo caduti nel burrone. Forse ce la facciamo. Forse riusciamo a fare ancora un passo indietro. Per fare questo, però, è necessario che tutti insieme realizziamo il superamento di ogni schema ideologico. Ce la faremo? Francamente, non lo so. Francamente, non sono convinto. La possibilità, però, ce la siamo data. La discussione continuerà ancora per giorni. Ho messo sul tavolo libri. Ho messo sul tavolo pubblicazioni. Sono a disposizione di tutti i colleghi che vogliano documentarsi anche meglio su questo. Vi prego, non votate questa proposta di legge come la voterebbe un *quisque de populo*. Approfondite ogni singola norma, anche chi è già convinto, in un senso o nell'altro, vada bene ad approfondire e a valutare ogni singola parola, perché stiamo decidendo di quello che sarà il futuro del nostro Paese. Marilena Grassadonia, dal palco del Pride,

e poi vorremo l'insegnamento *gender* nelle scuole. Tutte cose che sono state dichiarate da un palco, davanti a parlamentari appartenenti a due schieramenti qui presenti che applaudivano. Ditecelo chiaramente, allora. Il progetto che avete in mente è questo? Se questo è il progetto che avete in mente, non vi seguiremo mai e faremo la guerra, qui dentro e là fuori,

Una società in cui non si può più dire che un uomo è maschio e una donna è femmina è una società che non ha più nulla da dire. Questo è quello che dobbiamo dire ai nostri giovani, questo è quello che dobbiamo dire ai nostri figli!

Signor Presidente, io sono indignata. Mi verrebbe da dire che sono addirittura annichilita, perché è ormai da mesi, non soltanto adesso e non solo ora in quest'Aula, che abbiamo ascoltato per l'ennesima volta una fila di fuoco di *fake news* che, nel tempo, martellando continuamente, attraverso giornali, televisione e dichiarazioni, anche nelle Aule delle più alte istituzioni hanno alzato una cortina di fumo tossica. Una cortina di fumo tossica, attraverso cui non si riesce più a vedere la verità. Non si vede più, innanzitutto, il testo di legge in discussione, ma soprattutto ha fatto sparire le persone: le persone di cui questa legge si occupa; le persone che sono nostri concittadini e concittadine che chiedono, che sanno, che da venticinque anni hanno bisogno di tutele. Ed hanno bisogno di tutele perché all'improvviso siamo diventati tutti non omofobi in questo Paese. Siamo diventati il Paese dove i *gay*, le lesbiche i *transgender* possono vivere nella realtà più meravigliosa del mondo e dell'Europa. Nessuno ha un problema con l'omosessualità, né qui dentro né fuori. È incredibile come non ce ne fossimo accorti prima e si ha anche la sfacciataggine di riportare solo i casi dell'OSCAD 30 all'anno, con lo stesso gioco che si è fatto per decenni sulla violenza domestica e sulla violenza contro le donne: "quelle denunciate sono talmente poche. Il problema non esiste". È la stessa cosa. Le persone non denunciano perché non hanno gli strumenti per poter essere tutelate; non denunciano perché non ha senso denunciare, se poi l'omotransfobia non viene riconosciuta a livello penale. Non denunciano poi perché, perché, denunciando, fanno *coming out* il più delle volte e a casa i nostri giovani ancora non possono dire di essere *gay*, lesbiche o *transgender* perché vengono sbattuti fuori di casa. Di questo io non ho sentito parlare in quest'Aula, perché è di questo che si sta discutendo, non dei casi riportati dalla Gran Bretagna in un trafiletto di qualche giornale misconosciuto. Vengono raccontate storie storie incredibili e vengono rappresentate come se fossero all'ordine del giorno. In Commissione giustizia noi abbiamo dovuto subire lo stesso trattamento: 170 audizioni rigorosamente contrarie a questa legge, riportate addirittura come le posizioni uniche, sia dei giuristi che dei femministi che del mondo LGBT.

e ciò che non viene detto è ugualmente una menzogna, perché le parole contano. Ho sentito il collega Pillon fare l'elenco, in maniera anche sarcastica e ironica, di tutte le possibili definizioni con cui il mondo LGBT descrive se stesso (54) e ne ha parlato con quel ghigno da presa in giro che è proprio quello che ha tenuto sotto scacco queste persone e il mondo LGBT. LGBT. Sì, le parole contano: quell'elenco, che può essere trovato risibile da qualcuno, indica la ricchezza della natura umana che voi non potrete mai sconfiggere per quanto vi appigliate alla vostra ideologia. La natura umana è multiforme e le forme sono tante e sono diverse. Non possono trovare albergo nella nostra cultura e nella nostra società solo due forme di natura umana, ma deve trovare albergo tutta la variegata ricchezza della stessa, cosa che finora si è negata e negare questo significa negare l'evidenza. Fino a poco tempo fa anche qui in Italia l'omosessualità era perseguitata a norma di legge. Oggi ci scopriamo invece tutti liberali e non omofobi, ma è una cosa incredibile, che non regge. Come dicevo all'inizio, la cortina fumogena di *fake news* ha nascosto le persone; non solo, ha anche stravolto la verità delle responsabilità.

e il MoVimento 5 Stelle hanno il dovere morale di discutere e trovare soluzioni: se continueranno ad arroccarsi, saranno responsabili davanti al Paese di questo fallimento.

età e la poligamia e l'incesto non saranno più un tabù? E invece di rimuovere da quella delicata posizione la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, una persona cioè che afferma che l'omosessualità è equiparabile al fare sesso con gli animali ed è equiparabile alla pedofilia, cosa fanno fanno i colleghi Salvini e Pillon? La sostengono: finalmente abbiamo una persona seria e competente a ricoprire questo ruolo in maniera coraggiosa. E con queste persone noi dovremmo cercare una mediazione per contrastare le discriminazioni contro l'omolesbobitransfobia? E poi ripeto, il MoVimento 5 Stelle è orgogliosamente l'autore di tutte le politiche attive contenute in questo disegno di legge. Soltanto il perseguimento penale era contenuto in tutti i disegni di legge, ma noi abbiamo voluto gli sportelli di ascolto e i centri rifugio; noi abbiamo voluto i famigerati percorsi nelle scuole che voi continuate a diffamare affermando il falso: poco fa la collega Malpezzi vi ha dimostrato, carte alla mano, che non c'è nessuna obbligatorietà nessuna obbligatorietà per i corsi al rispetto e non all'educazione sessuale. E voi continuate invece a diffondere le vostre menzogne sulla pelle delle persone. Questo dibattito, che si è fatto così aspro e ideologicamente così insensato, si sta ripercuotendo sulla comunità LGBT, perché le aggressioni, gli attacchi, le discriminazioni e gli atti di bullismo sono aumentati. Ma voi siete ciechi voi siete ciechi perché non avete visto - fate finta di non aver visto - le piazze piene di persone, non solo di persone LGBT, ma della società civile. Da Roma, Milano, Torino, Palermo, Napoli, da ovunque

la legge di modifica costituzionale per abbassare l'età per l'elettorato attivo al Senato: adesso anche i diciottenni potranno votarci. Diamogli un motivo per appassionarsi alla politica, perché questo non è uno spettacolo dignitoso e non è uno spettacolo a cui i giovani possono guardare come esempio.

del collega Pillon - da esperto bibliofilo dovrebbe saperlo bene - portano le cose fuori dal buio: *fiat lux*. Le cose vanno chiamate col proprio nome e non bisogna metterci sopra una pecetta perché non le si vuole chiamare con il proprio nome. Le persone hanno stentato anche a riconoscersi perché non avevano le parole per definirsi. È ora che questo finisca e che tutte le persone possano essere libere di essere se stesse. Concludo dicendo che si può essere omofobi sia se si è analfabeti e illetterati, ma anche se si hanno tre lauree in più. L'illustre giurista che viene citato in quest'Aula come faro rispetto alle criticità di questa legge, il presidente Flick, è lo stesso giurista che ha affermato che l'orientamento sessuale è un fatto privato e che il legislatore non dovrebbe entrare nel merito. L'orientamento sessuale è un fatto sociale: è proprio questo che afferma il disegno legge in discussione; l'identità di genere è un fatto sociale. Ed è questo che la destra non può accettare: la legittimazione sociale delle diverse nature italiane. Ed è per questo che noi, invece, continueremo a sostenere questo disegno di legge e non accetteremo mediazioni al ribasso sulla

dare a Cesare quel che è di Cesare e dare al "sen" Malpezzi e al "sen" Licheri - così non si sentiranno offesi dall'aggettivazione di genere - e dare ai loro partiti, il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle, la paternità assoluta che rivendicano di questo disegno di legge. Gli italiani devono saperlo. Devono sapere che questa legge vi appartiene, cari colleghi.

legge. Nel momento in cui il nostro Paese è in preda a una grave crisi sanitaria ed economica, nel momento in cui, signor Presidente, resilienza che - non dimentichiamolo - ci indebita per centinaia di miliardi e che però necessità di tempi ristretti di riforme, di sblocchi delle procedure, imprese che attendono provvedimenti per uscire dalla crisi, nel mentre non riuscite a far altro che bloccare licenziamenti perché sul piano delle politiche attive ancora ieri, nel confronto con le parti economiche, non avevate una bozza di proposta reale, nel mentre bloccate gli sfratti perché non siete in grado di fare politiche sociali per la casa, nel mentre siamo nella piena crisi sanitaria e pandemica, nella piena crisi economica, nel mentre si parla della quarta ondata e quindi non ci sono ancora misure per rispondere al problema della scuola o dei trasporti, nel mentre il Paese soffre per questi problemi,

dopo lo *ius soli*, lo sbarco libero, la tassa di successione, non aspettiamo altro che il segretario Letta e gli alleati del MoVimento 5 Stelle, che su questi temi viaggiano spesso assieme, continuino su questa strada, ma ogni giorno gli italiani vi stanno rispondendo bocciandovi in tutti i sondaggi e in tutte le verifiche che vengono fatte.

di avere introdotto, come ha ben spiegato il collega Balboni ieri, il diritto penale dello stato d'animo interiore, cioè, un diritto penale - per chi capisce di diritto che è stato applicato solamente nel regime nazionalsocialista e in quello delle repubbliche sovietiche comuniste. Questa è la vostra legge di libertà.

vi rendete conto che state andando a colpire le libertà liberali, i valori liberali, i valori democratici, la libertà di pensiero, cari colleghi? State tranquilli che questa legge

il mio concetto di famiglia naturale, il fatto che ritengo un abominio l'utero in affitto, è evidente, è *in* *re ipsa* che in quel momento creo discriminazione. È ovvio che nel momento in cui sostengo che l'utero in affitto è un abominio e che la famiglia deve essere quella naturale di un uomo e una donna, in quel momento creo potenzialmente discriminazione, quindi sono passibile di condanna in base al codice penale. Questa è la realtà dei fatti, cari colleghi, altro che libertà e diritti; voi non state creando diritti, voi state sopprimendo diritti e, quel che è peggio, sopprimete i diritti del libero pensiero, andando contro la religione. Non per nulla la religione cattolica, come quella islamica, hanno espresso il proprio forte rammarico e la propria protesta. State violando, come espresso dal collega Malan questa mattina, le regole concordatarie; state violando ogni diritto per imporre la legge del pensiero unico. Voi volete imporre la comunità LGBT, ignorando i diritti degli altri cittadini, dei cattolici, dei religiosi, dei liberali, di coloro che credono e che non credono, ma che vogliono continuare a a poter esprimere liberamente il proprio pensiero senza essere tacciati da voi e dalla magistratura ed essere quindi incriminati e magari anche condannati fino a quattro anni di galera. Cari colleghi, zittire gli avversari con la galera è proprio è proprio dei regimi autoritari; è in Cina ed era a Cuba che si operava così e certamente anche nei regimi nazisti, dove vigeva infatti quel diritto penale penale dello stato d'animo interiore che prima citavo. Ecco dove volete portare il Paese. Ecco perché, cari colleghi, come ho detto all'inizio del mio intervento,

ha detto che non c'è nulla nell'articolo 7 e che nelle scuole non verrà fatto nulla. Allora, scusate, perché l'avete inserito? Perché avete inserito la giornata sul *gender*? Perché avete inserito l'articolo 7, se tanto non serve a niente? Invece basta leggere le cose e si capisce benissimo che voi nelle scuole di ogni ordine e grado - gli italiani lo devono sapere; ogni ordine e grado vuol dire, come il sindaco, senatore De Carlo, può confermare, dalla scuola dell'infanzia in avanti - volete andare a parlare del *gender*. Dovete spiegare che per parlare del rispetto di un qualche cosa, bisognerà pure spiegare cosa è quel qualcosa. Quindi voi dovrete spiegare al bambino di cinque anni cosa è il sesso binario,

che strenuamente si stanno battendo e hanno votato compatti, tutti presenti anche prima, la questione sospensiva, vorremmo continuare a poter parlare di mamma e papà, vorremmo continuare a poter dire che l'utero in affitto è una vergogna, vorremmo continuare a poter dire che i genitori non sono il genitore uno e il genitore due, ma la mamma e il papà. Continueremo, siamo certi che ce la faremo, siamo certi che questo testo liberticida, vergognoso e degno di uno Stato autoritario non verrà approvato da quest'Assemblea.

da molto tempo sentiamo il variegato mondo dei sostenitori del disegno di legge Zan raccontare in Aula, in televisione, in giro che il testo serve a ribadire la libertà individuale e sessuale di ognuno e a combattere contro le discriminazioni e le violenze contro gli omosessuali. ci sono quelli buoni e inclusivi, dall'altra parte i cattivi e gli omofobi. Questa è una menzogna, una delle tante menzogne tipiche della sinistra. Chiunque ci conosce, chiunque conosce Fratelli d'Italia, con il suo presidente Giorgia Meloni, sa bene che non c'è nessuno meno bigotto di noi, nessuno più inclusivo di noi e che nessuno di noi si sognerebbe mai di favorire qualcosa che possa andare contro la libertà individuale di qualcuno o contro gli omosessuali. Anzi, desidero dire che noi apparteniamo a una tradizione nella quale riconosciamo il valore del coraggio e oggi ci vuole grande coraggio a dichiararsi omosessuale *(Applausi)*, per di più a esprimere il proprio sentimento di amore nei confronti di una persona dello stesso sesso; c'è quindi tutta la nostra vicinanza nei confronti di queste persone

Quale libertà sessuale vuole difendere la sinistra? Penso alla stessa sinistra che ha l'abitudine di fare la morale, a comportarsi da censore, a guardare dal buco della serratura cosa fanno gli italiani, con chi fanno sesso, con chi si accoppiano, con chi vanno a cena. Ricordiamo le accuse a Berlusconi per le cene eleganti: quello non si poteva fare, la sinistra aveva deciso che era immorale.

il problema dei rapporti con quegli Stati che reputano l'omosessualità un reato penale. Invito i colleghi e i giornalisti che adesso stanno seguendo questi temi ad andarsi a rivedere gli atti di quel dibattito. Eravamo intervenuti quasi tutti (ricordo il senatore Balboni e io stesso); siamo chiesti come potevamo fare un accordo bilaterale con il Qatar, dicendo che dovevamo mandare le nostre scolaresche e i nostri ragazzi universitari a fare gli scambi culturali in Qatar, dove l'omosessualità è un reato penale, punito con il carcere e in teoria punibile con la pena di morte. Non ha senso. Abbiamo posto con forza questo problema, siamo stati gli unici in tutto il Parlamento a votare contro l'accordo bilaterale con il Qatar.

le loro foto da Dubai, dagli Emirati Arabi Uniti, dove l'omosessualità è reato penale, ma quando si tratta di fare soldi ce ne freghiamo dei diritti degli omosessuali

forse perché l'ex segretario del PD viene pagato dall'Arabia Saudita per parlare del nuovo rinascimento saudita e forse perché l'attuale segretario del PD

Intanto vorrei recuperare tutti i minuti che mi ha fatto perdere. PRESIDENTE. Non ne ha persi molti e, come sempre, il tempo che viene impiegato nelle interruzioni viene recuperato. Stia assolutamente tranquillo su questo, non è un'innovazione nei suoi confronti. FAZZOLARI *(FdI)*. Confido che non mi toglierà la parola quando sentirà qualcos'altro che non le piace. Se vuole le fonti, l'editoriale «Domani», che non pare essere particolarmente vicino a Fratelli d'Italia, è quello che riporta in modo puntuale queste informazioni sugli

100.000 euro l'anno per otto sedute presso lo stesso gruppo societario che cura l'immagine della casa saudita. Ecco perché non si parla degli omosessuali condannati a morte in Arabia Saudita. Si parla invece della legge ungherese che vieta la propaganda *gender* nelle scuole. Perché? Perché Orbán non stacca gli assegni che staccano i qatarioti e i sauditi ai politici italiani ed europei: ecco perché. C'è una mozione di Fratelli d'Italia al Senato e alla Camera per chiedere di condannare i Paesi nei quali l'omosessualità è reato: l'ha presentata Fratelli d'Italia (nessun'altra forza politica l'ha presentata), perché noi siamo persone libere che hanno la forza di dire chiaramente come stanno le cose e di condannare là dove la violenza contro gli omosessuali è vera e concreta. Le altre forze politiche invece si esimono da questi atti di coraggio. Il perché lo sappiamo. di legge Zan decide che il sesso biologico non esiste, esiste invece l'identificazione percepita di sé. Vuol dire che se mi sento donna, sono donna e se vado da qualcuno a dire che sono donna e lui insiste che sono uomo lo posso denunciare per discriminazione.

Chi sostiene queste cose dovrebbe giustificare le idiozie che dice. Abbiamo degli esempi su che cosa succede quando si decide che il sesso è autopercezione. In Canada, dove già c'è la legge Zan canadese, un attivista trans, nato uomo che adesso si dichiara donna, ma non è operato, Jessica Yaniv, ha l'abitudine di andare nei centri estetici femminili e chiedere alle estetiste di depilargli i genitali, ovviamente maschili, e chi si rifiuta viene denunciata per Chissà quanti burloni in Italia, se dovesse passare la legge Zan, decideranno per mezz'ora di dichiararsi donna chiedendo a qualche ragazzetta estetista gli depilargli le parti intime. Poi abbiamo gli esempi dello sport, che sono gli stessi: gli Zan di tutto il mondo hanno deciso che se uno si dichiara donna partecipa alle competizioni femminili e non con gli uomini. Alcuni esempi:

Maxine Blythin, giocatrice transgender di cricket: quando gareggiava con gli uomini aveva 15 punti segnati al lanciatore (ottima media), adesso la sua media è 123 (addio sogni di gloria alle lottatrici avversarie). Lauren Hubbard sarà la prima *transgender* a partecipare alle Olimpiadi nel sollevamento pesi e ovviamente le sue avversarie non l'hanno presa benissimo. È anche un problema di sicurezza sono alcuni esempi concreti: la federazione gallese di *rugby* ammette i giocatori transessuali, dall'anno prossimo anche quella francese. Un esempio: Kelly Morgan. Si legge, nei resoconti di una partita, che ha piegato la sua avversaria come una sedia a sdraio, con fratture multiple. Ma vogliamo vogliamo togliere la gioia a Kelly Morgan di giocare con le donne, se si sente donna? Ma c'è di meglio. Fallon Fox è un lottatore o lottatrice di arti marziali miste (MMA per chi lo conosce), lo sport più violento che ci sia; si sente donna e combatte contro le donne. Alcuni commenti: Fox, un atleta maschio *transgender*, ha distrutto Erika Newsome in un combattimento MMA in Florida, durante il quale ha assestato un colpo alla testa con il ginocchio mentre la teneva ferma con le mani, lasciandola priva di sensi. Per l'esattezza, le ha spaccato il cranio. Queste invece le dichiarazioni di Tamikka Brents, un'altra sua avversaria che è uscita dall'incontro con sette fratture facciali e una commozione celebrale: «Ho combattuto contro molte donne, mai avevo avvertito la forza e la ferocia che ho sperimentato quella sera con Fox, e sono una donna forte. Continuo a disapprovare che Fox combatta contro le donne; lo trovo ingiusto e non leale». veramente pensate che queste siano parole omofobe? Ma vi rendete conto della follia cui siamo arrivati con la furia ideologica che avete? E certo che le femministe sono contro di legge Zan, perché vorrebbero difendere le donne, che rischiano di uscire con le ossa rotte da questa legge, sul *ring*, quando devono combattere in combattimenti come questi, e nella società, quando si vedranno private dei loro diritti. giusto combattere ogni discriminazione e violenza contro le persone omosessuali; su questo avreste il pieno appoggio di Fratelli d'Italia. Ma non è questo che fa il testo di legge Zan, che è un testo ideologico, liberticida, pericoloso e che discrimina le donne. Per questo piace alla sinistra e per questo gli uomini e le donne libere la combattono.

dispiace che non ci sia il senatore Bressa, che quest'oggi ha cercato di fare una ricognizione nell'ambito dell'ordinamento, individuando le norme che richiamano il concetto di identità di genere sia nella nostra legislazione che in quella europea o comunque nella legislazione dal punto di vista generale.

sostenere che l'identità di genere e quindi il diritto all'autodeterminazione del genere siano un principio costituzionale. Si dimentica tuttavia di dire che quella è una sentenza interpretativa

nodale importante, perché diversamente passa l'idea secondo la quale l'identità di genere, che è una sovrastruttura una sovrastruttura (cioè l'idea secondo la quale io devo essere riconosciuto per come percepisco me stesso), sia di per sé un diritto assoluto, valido *erga omnes*. omnes*. Non mi pare che sia così e non mi pare che la sentenza di riferimento del 2015 dica questo. e del dibattito che si è tenuto all'interno e fuori dalle Aule parlamentari, nei giornali e nelle varie riviste, molti giuristi, che qui non sto ad indicare per ragioni di brevità, hanno

porta con sé delle dubbie valutazioni sulla portata effettiva di alcune norme. Si è deciso, alla Camera dei deputati, di inserire le fattispecie della discriminazione e dell'istigazione alla discriminazione per motivi

viene meno il principio di tassatività della norma, essendo assolutamente indeterminata la fattispecie. Sappiamo infatti che il reato, per definizione, è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Questo di fatto comporta che si lasci al giudice la valutazione di ciò che è discriminatorio e di ciò che non lo è. Mi permetto di dire che l'ubiquità del termine discriminazione è anche discernimento e il discernimento vuol dire scegliere, valutare ed esprimere un'opinione. Nel concetto stesso della discriminazione c'è il riferimento all'opinione e alla valutazione che ciascuno può avere nell'affrontare nell'affrontare un determinato aspetto e un determinato problema. una parte dello schieramento, che propugna l'applicazione del disegno di legge Zan così com'è, compie un errore dal punto di vista politico e strategico. Non si può accettare che un tema di questa portata sia di fatto ridotto ad una prova muscolare. Questa non è politica e non è il servizio che il Parlamento deve fare rispetto a presunti diritti, che ritenete siano stati o vengano violati oggigiorno. Consentitemi

dicitura è la conseguenza di un compromesso raggiunto tra le diverse forze politiche, nell'ambito della discussione alla Camera Al di là di questo, è chiaro che il riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione, non solo è pleonastico, perché comunque il principio costituzionale esiste al di là di ciò che scrive la norma, ma è anche controproducente, perché la parte finale dell'articolo 4 porta a considerare e a far rientrare nell'alveo penale determinati comportamenti che forse non hanno alcuna

complicate, tipo quella sull'identità di genere, che appartiene ad un concetto che è la sovrastruttura ideale e idealista

che contiene in sé il diverso e una molteplicità di aspetti, non la separatezza, né ciò che volete difendere e di fatto discriminate. La dichiarazione dell'universalità degli uomini e della loro uguaglianza contiene in sé tutte quelle definizioni che pensate invece di voler inserire, ipostatizzandole all'interno di una norma la cui portata è contraria alle sue premesse. Qualcuno la chiama

nel concetto di ciò che doveva essere una minoranza e finisce per avvertirsi o per essere riconosciuto come un aspetto qualificante, di una portata

Inviterei l'Assemblea a riflettere su questo aspetto, perché ritengo che nel concetto di uomo e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ci stia tutto:

Non ritengo che tutto debba essere buttato al macero: sicuramente il dibattito in Parlamento ha prodotto

Signor Presidente, esordirò anch'io, come il senatore Dal Mas, con un fastidio e un dispiacere, che è quello di vedere gli scranni vuoti, in effetti, a partire da quelli di coloro che sul tema si dicono più accalorati e che poi vengono anche in Aula a fare dimostrazioni molto di peso, come direbbero loro. Nella realtà dei fatti, di peso ne abbiamo sentito poco anche negli interventi. Si è visto più, invece, un atteggiamento che a me non piace e che definirei fazioso, provocatorio, tignoso, rigido, per nulla

rispetto alle cose che si vogliono fare, perché è come dire che chi vuol essere tollerante ammette qualsiasi cosa che corrisponda al proprio pensiero, ma, quando non corrisponde al proprio pensiero, esclude qualsiasi possibilità di accordo. Questa non è tolleranza, ma arroganza, che è un'altra cosa.

fondamentale cui qualsiasi cosa votiamo in quest'Aula dev'essere sempre improntata. Quando siamo al Governo, siamo tolleranti e rispettiamo, siamo liberali e accogliamo le idee degli altri. Sappiamo che a una parte di sinistra questi concetti sono estranei:

Quindi, si fa un po' fatica a vedere questa esacerbazione delle espressioni come se fossimo in un Paese tribale, nel quale si sta iniziando a mettere qualche piccolo tassello di legge per imporre il rispetto delle altre persone. Non è così. L'altro giorno mi sono trovato in un dibattito nel quale la controparte argomentava che serve approvare il disegno di legge Zan così com'è, parola per parola, per impedire che ci siano ancora omosessuali, transessuali o altri picchiati per le strade. Cosa stiamo dicendo? Per le strade non dev'essere picchiato nessuno. Non è che se sei di una categoria, se sei interista o milanista, hai diritto a non essere picchiato e, se sei juventino, devi esserlo. Non è che, se sei bianco, puoi essere indenne dalle botte e, se sei nero, devi essere picchiato. Cosa stiamo dicendo? Questo tipo di categorie non può esistere in un Paese civile. Tutti hanno il diritto di essere liberi e tutelati. *(Applausi)*. Il paradosso cui stiamo arrivando è mettere categorie che non sono privilegiate, ma è come se fossero quasi protette. che ci siano categorie che hanno meno diritto a essere tutelate rispetto alla discriminazione. No, la discriminazione non deve esistere nei confronti di alcuno, parlando ovviamente in termini positivi. L'abbiamo detto e lo stiamo dicendo in tutti i modi: troviamo un'intensa. Ci è stato opposto un argomento: poiché in Commissione il disegno di legge è rimasto per nove mesi, evidentemente non c'è la volontà di arrivare a un'intesa. Presidente, nelle Commissioni del Senato, come in quelle della Camera, ci sono disegni di legge su qualsiasi argomento, dall'handicap fino ad arrivare all'economia, dalle tasse ai diritti sociali, che dall'inizio della legislatura sono in attesa di essere mandati nelle Aule ed essere dibattuti. Penso a quello sui *caregiver*, per avere un esempio. Il disegno di legge presentato dal sottoscritto era il n. 7 della legislatura e mutua da quello fatto dalla senatrice Bignami in quella precedente: non è neppure stato abbinato, tanto per avere un'idea. un'idea. Non argomentiamo in maniera faziosa, ma diciamo invece in maniera molto corretta che, se c'è una volontà politica, le cose si fanno. Un adagio dice che la politica è l'arte di rendere rotondo ciò che è quadrato: tutto si può fare, basta volerlo. È evidente che, se nei nove mesi passati non si è trovata un'intesa, è perché non c'era la volontà di trovarla, da una parte e dall'altra. Può essere. Certamente dichiariamo - e lo stiamo dicendo in tutti i modi - di essere disponibili a cercare un'intesa sul merito dei fatti. Può essere fatto nelle prossime due settimane? Abbiamo visto questa mattina respinta la questione sospensiva in questo senso, ma può essere fatto ancora, arrivando a una stesura di emendamenti condivisa. Certo che sì. Credo che sia da cogliere

quel solo voto di scarto significa che si sta portando avanti qualcosa di divisivo, che non ha avuto la capacità e non è stato improntato per mettere assieme e riunire. e riunire. A questo punto, è evidente che l'obiettivo è solo quello di mettere una bandierina politica, ideologica, che nulla ha a che fare col merito. Su questo devo riconoscere una grande capacità mediatica di certa parte della sinistra nel vendere i titoli. Vedo il senatore Cangini che mi ricorda i giornali, come a indicare chi vende i titoli sui giornali, senza guardare a ciò che è scritto nell'articolo stesso. C'è chi è capace di farlo e qualche giornale mette addirittura le fotografie e tutto il resto sotto, in secondo piano. Presidente, abbiamo bisogno invece di parlare del merito. Il presidente Ostellari ha dato un'eccezionale dimostrazione di buona volontà e di pragmatismo. Ecco, partiamo da quegli elementi. Ne cito solo uno, l'articolo 4, che dovrebbe essere un presupposto di pluralismo e recita appunto: «Pluralismo delle idee e libertà delle scelte»; «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Signor Presidente, immagini adesso che un cittadino all'esterno, ascoltando il mio discorso, che ritengo improntato a una significativa pacatezza, vada poi al compiere gesti estremi di intolleranza; tranquillamente, seguendo questo percorso, un magistrato potrebbe chiamarmi a rispondere, ritenendo che abbia istigato quella persona a commettere un atto di violenza, pur essendo totalmente disgiunto il fatto

Nel momento in cui si mette nelle mani di un magistrato la scelta se una tale affermazione possa essere foriera di atti di odio o di istigazione all'odio, ripercorriamo strade che abbiamo già visto distorte, poi, all'interno dei tribunali, per le quali alla fine una persona, che nulla ha a che fare con un atto di violenza, per questioni politiche viene chiamata a rispondere in tribunale.

Questo significa comprimere i diritti. Stiamo dicendo in tutti i modi, signor Presidente, che c'è ancora tempo e ancora spazio per trovare un'intesa; bisogna trovarla altrimenti è evidente che al Partito Democratico e a certe ali estreme della sinistra interessa semplicemente piantare una bandierina, andando poi, con ciò, ad aprire falle significative nella tutela della libertà delle persone, di tutte le persone, signor Presidente, senza alcuna distinzione di sesso e di genere. Perché la libertà o appartiene a tutti o è una negazione che va a subire chiunque di noi.

sono passati tanti mesi da quando in quest'Aula, sui *social* e sui giornali abbiamo sentito le dichiarazioni di chi si apprestava a supportare il nuovo-vecchio Governo,

avrebbe imposto subito una riflessione, sul salvarla da chi: da chi l'aveva portata fino a quel punto e cioè dagli stessi che si proponevano, poi, di salvarla; questo, però, è un altro tema. *(Applausi)*. perché oggi quegli stessi che si proponevano di salvare la nazione, anziché occuparsi di una pluralità di persone prive di diritti, come quelli economici (perché a tanti i ristori devono ancora arrivare), dibattono di una questione diventata importante perché qualcuno si è accorto di quanto sia liberticida, mentre fuori c'è gente che non ha ancora ricevuto i rimborsi per la situazione gravissima che ha patito durante il *lockdown*. *(Applausi)*. Questo bisogna che sia chiaro, altrimenti tutta la discussione che facciamo, indipendentemente dalle rispettive posizioni,

in qualche maniera, supportata da un Governo che doveva salvare la nazione.

fuori, in condizioni difficili, questa nazione ha cercato di risollevarsi, dentro ci occupiamo di limitare la libertà degli unici che dissentono anche sul vostro atteggiamento nei confronti dell'economia e della parte produttiva di questo Paese. Quindi, c'è una doppia

per piantare una bandierina, per far credere a qualcuno di essere rappresentativi ancora di qualcosa. Credete, nella vostra assoluta autoreferenzialità, di rappresentare qualcuno. In realtà, rappresentate, male, una minoranza di persone che, invece, guarda caso, ha più necessità di interventi sulla parte economica in questo momento, perché sulla parte giuridica si sente già tutelata da leggi già esistenti, dal codice penale, da un atteggiamento

o ce ne sono ben poche, a dimostrazione anche della percezione della paura di certe minoranze, che io faccio fatica a definire minoranze. Ma perché, infatti, dobbiamo ghettizzare le persone? Perché dobbiamo dividere le persone tra quelle che hanno un orientamento sessuale come il mio e quelle che hanno un orientamento sessuale differente? Noi Noi di destra siamo sempre stati diversisti quando voi volevate appiattire tutto e omologare il mondo come nell'ex Unione Sovietica. Ma non siamo diversisti sui diritti. Per noi tutti hanno gli stessi diritti e non abbiamo bisogno di trincerarli all'interno di una ricostruzione della società fatta da voi a vostro uso e consumo. Noi crediamo che il cittadino non sia solo LGBT o non LGBT, ma sia cittadino nella pienezza dei suoi diritti, che è anche il diritto di poter dire la propria opinione quando non si condivide quello che voi vorreste si dicesse. abbiano la possibilità di emanciparsi anche sotto il profilo del lavoro e non di restare schiavi vostri, con il reddito di cittadinanza che avete istituito per avere persone sempre a vostra disposizione. Questo vorremmo. Vorremmo ampliare i diritti, non limitarli. Invece voi, con questa legge, li limitate fortemente. Anzi, peggio ancora: limitate i diritti di coloro i quali non la pensano come voi, credendo che si debba, in qualche maniera, discriminare il pensiero diverso dal vostro. Ancora una volta, discriminate il diverso; ancora una volta, lo chiudete in un ghetto; ancora una volta, gli togliete il patentino. Chissà, poi, perché voi. Chissà, poi, perché voi potete consegnare a qualcuno i patentini. Dall'alto di cosa? Qual è la ragione che vi dà la facoltà di dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Da cosa vi deriva? Dal consenso popolare? Insomma, fatevene una ragione, perché non mi pare proprio. Dal fatto che voi avete una superiorità culturale? Anche questa convinzione dovrà cadere, perché io, quando vedo professori che incitano all'odio, rovesciando i libri della Meloni in una

il dominio di questa società e sta accadendo perché state perdendo il consenso, perché non siete neanche più rappresentativi dei mondi che fino ad ora vi hanno consentito di sedere qua dentro e non parlo neanche più degli operai, perché ormai li avete dimenticati da anni, quelli puzzano, così come avete dimenticato i contadini, che lavorano e si sporcano le mani. Sono tutte cose talmente diverse dai vostri salottini *radical chic* che non potete comprenderle, tant'è vero che vincete nei centri storici e perdete in tutte le periferie perché non rappresentate nemmeno più la visione di quello che era il vostro bacino elettorale. Che cosa fate allora? Cercate di cancellare quelli che rappresentano la vostra alternativa; lo fate cercando di zittirli, dicendogli che non possono parlare perché, non solo hanno un'idea diversa dalla vostra, ma hanno un'idea che che per giudizio vostro - e quindi divino - non può neanche permettersi di essere rappresentata. Questi siete voi, questo è lo scopo di questa legge: tapparci la bocca semplicemente perché sapete che, se noi parliamo o continuiamo a farlo, la vostra stessa esistenza viene meno. infatti diceva un vecchio adagio, se non ci fossero i brutti, non si vedrebbero i belli. Ecco, voi cercate di cancellare i belli per sembrare belli voi; in realtà rimanete brutti, come la politica che avete fatto in questi anni, come l'imbruttimento delle istituzioni che avete cercato di fare

non hanno una crisi di coscienza; hanno semplicemente acceso la coscienza, rendendosi conto che quelli fuori, le persone che gli hanno sempre dato fiducia non vogliono che si occupino di questa cosa; vogliono che vi occupiate di economia, economia, che estendiate i diritti a tutti e non li ghettizziate in un angolo, facendoli sentire ancora diversi. A me danno fastidio i locali solo per i *gay* o solo per le lesbiche. Io credo che i locali debbano essere sempre per tutti: non c'è un'*apartheid* nei confronti di qualcuno; ognuno deve essere libero di andare nel locale che vuole. Il ghetto fa parte di un'altra cultura, di un altro sistema di vedere la società. Noi siamo diversi, continueremo a dirlo finché avremo voce, finché gli strumenti anche del dibattito parlamentare ce lo consentiranno e fino a che anche nelle piazze potremo andare a spiegare veramente che cos'è il disegno di legge Zan, al di là del vostro *storytelling*, della vostra narrazione di parte, che ogni qualvolta si fa un dibattito pubblico poi si scioglie come neve al sole. Continueremo ad andare nelle piazze a dirlo e non sarà in discussione - a impedirci di farlo e non sarete certo voi, che ormai rappresentate poco più che una minoranza, a dirci quello che dovremo fare e quello che dovranno fare gli italiani. *(Applausi)*.

prima di fare il mio intervento vorrei formulare delle domande che mi sono posta in questi giorni e che vorrei condividere con voi. Siamo certi che questa proposta di legge sia necessaria e sufficiente ad assicurare la lotta all'odio e l'accettazione di quelle categorie che si intende tutelare? Il termine «categorie» non è una scelta casuale ovviamente, perché questo stiamo realmente creando. Può un'imposizione normativa determinare un cambiamento culturale e comportamentale? Nell'articolo 4 non si parla, ad esempio, né di dignità né di persone; in realtà, in questo modo affrontare il tema come un pensiero ingabbiato dal penale. Ma un pensiero di questo tipo può portare al bene? Allora mi sono venute in mente alcune esperienze del passato legate in particolare allo studio del testo di un autore, Gary Chapman, che è un

abbiamo scelto e che ci sta accanto, ma siamo certi di amarla nella misura in cui lei desidera essere amata? Dove voglio arrivare con questo? Voglio dire: siamo certi che questo provvedimento normativo intervenga a

dedicata all'omolesbobitransfobia, cosa si propone? Si riconosce «il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro lo omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni, le violenze» e quant'altro (per noi è tutto noto). Arriviamo al comma 3 dello stesso articolo: «In occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri» - attenzione a questo punto - «e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1». «Le scuole, nel rispetto del piano triennale» - quindi il PTOF - «dell'offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

tra le parti, quindi al momento dell'iscrizione dei ragazzi a scuola tra la famiglia e la scuola. In quanto tali, si tratta di progettualità di massima. Sappiamo benissimo che poi *in itinere,* nell'arco di tre anni, vengono poi proposti dei progetti *ad hoc*, in base anche all'esigenza formativa determinata proprio dalla libertà didattica di insegnamento del docente stesso. stesso. Da questo punto di vista, ritengo che ad esempio ci sia un problema non indifferente che riguarda la liberatoria. In questo In questo modo noi cosa faremmo? Daremmo libertà assolutamente alla scuola, chiaramente previa firma e sottoscrizione da parte dei genitori, di poter mettere in atto un'attività formativa verso una certa direzione. Tuttavia, per conoscere nello specifico e precipuamente i progetti proposti annualmente, è opportuno che le famiglie sottoscrivano una liberatoria

negli articoli 1, 7, 9, 10; non vi sono riferimenti specifici, anche quando addirittura si parla di centri nell'articolo 9.

Io sono stato il primo non vedente al Governo, ho chiesto all'INPS quante sono le persone con disabilità. Siamo 7,5 milioni, prima c'era una stima! Dei nostri problemi non ce n'è traccia nel *recovery*, la legge 112 sul dopo di noi è sottofinanziata, mancano i decreti attuativi della legge sui *caregiver* - i familiari costretti a prendersi cura del parente - per stanziare i fondi e disciplinarne il regolamento di attuazione, anche sul fronte previdenziale, ci sono sette proposte diverse al Senato sul tema, altro che ddl Zan. La pensione di invalidità è di 285 euro, grazie a una sentenza della Suprema corte per talune categorie è salita a 600 euro. E nessuno ne parla». si parlava anche della dimensione della sessualità per le persone con disabilità. Cosa mi preme evidenziare? In questi mesi abbiamo assistito

ripeto, quella sinistra di cui prima facevo parte e che, proprio dall'esperienza che ho vissuto anche in riferimento a questo disegno di legge, ha suscitato in me l'esigenza non di passare dalla porta accanto ma di fare il salto, come dico spesso, della barricata. Voglio segnalare che assistiamo a un'ingerenza anche governativa sul tema oggetto del disegno di legge Zan. Mesi fa è stato fatto un corso di aggiornamento per le Forze dell'ordine, durante il quale sono state affrontate le tematiche di interesse generale per l'anno 2021. La seconda giornata portava il titolo «Quando l'odio diventa reato» con riferimento alle discriminazioni, portando ad esempio situazioni legate all'orientamento sessuale. Si fa spesso riferimento - all'interno del corso di formazione - a una *vacatio legis*. Concludo portando un altro esempio di ingerenza governativa a cui abbiamo assistito anche ieri, quando, al di là della persona che stimo profondamente, durante d'Assemblea, anche la Sottosegretaria all'istruzione ha pubblicato su Facebook un suo *post* facendo riferimento all'articolo 7 e indicando una prospettiva che si vorrebbe auspicare rispetto all'articolo 7, ma non il contenuto dello stesso. Quindi, da questo punto di vista, se da un lato, attraverso produzioni cinematografiche, *talk-show* e addirittura cartoni animati per bambini, si è cercato di

di legislatura, i miei primi tre anni di legislatura, prendo la parola in quest'Aula scosso da un timore e chi mi conosce sa quanto poco sia timoroso nel difendere o nell'esprimere le mie posizioni. Il timore è quello di essere equivocato o peggio di essere proscritto dal consesso civile e considerato persona mostruosa. Mi conferma e mi conforta il fatto che tesi analoghe a quelle che andrò ad illustrare sono state in questi giorni espresse da illustri costituzionalisti, giornalisti, intellettuali personalità politiche tutte di sinistra e, quindi, forse il marchio di infamia ricadrà con debolezza su di me e su di loro. Il problema c'è e credo che

coerente con lo spirito dei tempi che ci è dato vivere. Coerente con il dilagare di un politicamente corretto eretto a dogma e con un processo sistematico di sradicamento e di sistematica perdita dell'identità delle persone e delle società. Coerente con una tendenza sempre più forte e - oserei dire - violenta non solo di riscrivere, ma addirittura di cancellare la storia su basi etiche.

su «Repubblica», proprio parlando del disegno di legge Zan - con la tendenza a far proliferare diritti che non hanno più nulla a che vedere con la società o con i cittadini intesi nel loro complesso, ma che si rivolgono a singoli gruppi sociali e a singoli gruppi di cittadini - scrive Ainis in chiave critica - i cui desideri vengono di conseguenza trasformati in norme in norme giuridiche. Colleghi, capisco che questo tutto questo nasca da una spinta positiva volta a fare del bene, a fare giustizia. Tutto questo però non ha davvero nulla, ma proprio nulla, di liberale. Credo e ho sempre creduto che i diritti delle minoranze sessuali o non sessuali - vadano sempre e comunque salvaguardati ed equiparati ai diritti della maggioranza, ma non per vezzo intellettuale, ma perché questo è quello che prescrive la Costituzione. All'articolo 3 della Costituzione è scritto che «Tutti i cittadini

Non meno importante dell'articolo 3 della Costituzione è però l'articolo 21, che prescrive che tutti hanno la libertà di esprimere le proprie opinioni. È un articolo che mal si concilia, per esempio, con il desiderio di imporre una certa visione del mondo, giusta o sbagliata che sia, o della natura umana ai giovani delle scuole. Non è così che si sanano i pregiudizi e che si rende giustizia a chi giustizia non l'ha avuta e riconosciuta. Io credo che il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni vada salvaguardato sempre e comunque soprattutto quando non si condividono le opinioni in questione e soprattutto quando quando le si giudichi mostruose. Vorrei e voglio che ciascuno di noi sia libero di dire che Hitler o Stalin siano stati i benefattori dell'umanità, piuttosto che dire che in natura non esiste l'omosessualità o, al contrario, che in natura non esistono i generi sessuali e che tutto è dovuto a condizionamenti sociali. Colleghi, le sciocchezze, i pregiudizi, le fesserie e le mostruosità intellettuali si commentano da soli e da soli si marginalizzano. I divieti non rafforzano, ma indeboliscono le giuste posizioni. A furia di aggiungere categorie a categorie e divieti a divieti, si fanno torti più che giustizie perché ogni categoria che aggiungiamo, per esempio, al novero delle categorie contemplate dalla cosiddetta legge Mancino ne esclude altre. So di dire una cosa non tollerabile nella temperie del clima che si è creato, ma io considero sbagliata e illiberale la legge Mancino e ritengo che ogni gruppo sociale o categoria o gusto sessuale viene ricompreso di volta in volta in quella legge crei un vuoto rispetto ad altri gruppi sociali e ad altre categorie e leda di fatto i diritti di altri gruppi sociali e di altre categorie. Faccio un esempio paradossale, ma fino a un certo punto: tutti quanti abbiamo ben chiaro quante e quali sofferenze un ragazzino sovrappeso deve sopportare nell'essere sistematicamente dileggiato dai propri compagni di scuola. Allora che facciamo? Mettiamo anche i ciccioni tra le categorie che la legge Mancino protegge *(Applausi)*? Davvero, perché no? Allora i portatori di occhiali, i cacciatori, i vegani, non c'è limite alle categorie umane e alla volontà di certe persone di annullarsi e identificarsi in un singolo aspetto particolare della propria vita. Non è questo però che fa di noi una società, non è questo che fa di noi dei cittadini di uno Stato. Più aggiungiamo, più escludiamo; più proteggiamo, più danneggiamo *(Applausi)*. Questo dovrebbe essere il concetto che dovremmo avere tutti quanti ben chiaro. Colleghi, stiamo esagerando, si sta esagerando, forse da entrambe le parti, ma si sta esagerando su questo tema e sul disegno di legge Zan. Io ho sentito in quest'Aula la collega Malpezzi,

dalla collega Malpezzi è che quel testo salva delle vite umane. È esagerato, è davvero esagerato, e se fosse vero vorrebbe dire che i Governi di Centrosinistra retti da maggioranze organiche di Centrosinistra si sono resi responsabili di morti.

Non è sensato ritenere che, in un contesto di larghe intese, una legge cara a una parte politica debba necessariamente essere approvata anche dall'altra parte politica, sapendo che questa è una legge discussa e discutibile. il sottoscritto e quel che resta del mio partito volessero a tutti i costi far passare una norma per la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e inquirente. È un principio che io condivido e che ritengo essenziale in termini di civiltà del diritto;

inastando una bandiera demagogica, indipendentemente dalla fine che farà il disegno di legge in questione. La demagogia è nemica della politica, che si regge sul compromesso, che non è una parolaccia. È una parola sprezzata da molti, da troppi probabilmente, ma è l'essenza della politica: nasce da un compromesso l'Unità d'Italia, nasce da un compromesso la Costituzione repubblicana; ogni norma che rispettiamo e di fronte alla quale ci inchiniamo, approvata da questo Parlamento in questa e nelle fasi storiche precedenti, è nata da un compromesso. Il compromesso viene negato dai demagoghi, dai despoti e dai moralisti, categorie personali e sociali che usano brandire la clava dell'etica per darla in testa a chi la pensa diversamente, facendo così dell'avversario un nemico, non della propria parte politica, ma della civiltà *(Applausi)*. Questa, colleghi del Partito Democratico, è la strada che avete imboccato ed evidentemente conduce ad un vicolo cieco. Allora, se non lo fate per ridare dignità alla politica, se non lo fate per dare agibilità alla vostra parte politica, se non lo fate per difendere i diritti che dite di voler difendere, fatelo per voi stessi. C'è solo una cosa da fare per salvare tutto questo: innestare la retromarcia *(Applausi)*.

da diversi mesi il tema del disegno di legge Zan tiene banco nei dibattiti televisivi, nelle piazze, nelle nostre caselle di posta elettronica. Siamo stati bombardati incessantemente da propaganda che pone in evidenza una sola versione dei fatti e una sola visione. I giornali e le televisioni si sono alternati nel dipingere tutti coloro che non sono a favore di questo disegno di legge come retrogradi, omofobi, razzisti (e chi più ne ha più ne metta), come se improvvisamente i diritti civili non facessero già parte della nostra società. È doveroso mettere ordine davanti a tanta demagogia, mettere ordine davanti a tanta demagogia, perché oggi ci troviamo a discutere un testo totalmente ideologizzato, voluto da chi pensa che debba prevalere tutto ciò che è minoritario, a discapito della maggioranza silenziosa.

Per questo parlo di elettorato disinformato. Alla Camera si è di fatto ritenuto che i principi della nostra Costituzione non andassero più bene e si è voluto approvare una legge che introduce la tutela di un concetto ideologico, quello del *gender,* distinto e sovrapposto a quello del sesso biologico. È un disegno di legge che vorrebbe introdurre sanzioni penali e persino pene accessorie, vale a dire rieducative, da scontare in istituzioni e associazioni che si occupano delle tematiche relative al disegno di legge per chiunque osi o sembri affermare che la natura è quella di maschio e femmina. legge che introduce una Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, in occasione della quale le scuole provvedono alle attività, anch'esse di promozione ed educative. Avete stanziato a favore delle associazioni LGBT quattro milioni di euro. Basterebbe informare correttamente gli italiani di queste vostre intenzioni per sollevare uno scontro ideologico senza precedenti ed è forse quello a cui state puntando. Attenzione, perché state dando vita ad un clima di scontro ideologico, che ha un inizio ma non ha una fine, e di questo siete responsabili. Se volessi essere provocatoria o ironica vorrei sapere cosa pensereste se vi fosse proposto di istituire anche una giornata contro l'eterofobia o per l'orgoglio etero. Chissà dove andremo a finire. Andiamo, per favore, a valutare le questioni serie e pratiche che interessano gli italiani e vi chiedo: il disegno di legge Zan potrà impedire o limitare molestie, insulti o violenze? Non necessariamente, perché il nostro codice penale già punisce insulti, molestie o violenze, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione o opinione politica. Vi voglio ricordare che la Lega ha già proposto di inasprire le pene che già ci sono, ma avete detto di no: anche questo dovete dire agli italiani. Il vostro disegno di legge servirà a dare diritti fondamentali alle persone omosessuali, trans, eccetera?

matrimonio. Diciamo agli italiani, compresi i vari *influencer* che tanto amano creare scontri ideologici, quali sono le conseguenze di questo disegno di legge così come scritto e proposto: impedire la libertà di parola, perché ogni posizione diversa potrebbe essere considerata un probabile incitamento alla discriminazione; cancellare i termini «padre» e «madre», sostituendoli con «genitore 1» e «genitore 2»;

che sposare un uomo o una donna è perfettamente uguale e che i bimbi nascono anche da due padri o da due madri. Si chiede da anni di insegnare l'intelligenza emotiva nelle scuole e noi rispondiamo istituendo un obbligo allucinante come questo.

che mirava a punire veramente le discriminazioni, modificando, come proposto, gli articoli 1, 4 e 7. Le vostre vere intenzioni sono altre. Oggi ci sono molti esempi di celebri coppie omosessuali che fanno figli attraverso l'utero in affitto; una volta approvata la legge, sarà facile accusare di discriminazione chi è contrario a tale pratica, che di fatto incoraggia la mercificazione di madri che portano avanti la gravidanza a uso e consumo della coppia di turno. Per molti anni della mia vita ho pensato che non avrei avuto dei figli. Ma, quando poi capita questa fortuna, comprendi che non stai soddisfacendo una tua necessità o un tuo egoismo; realizzi che si tratta di un dono della natura. E non ho mai pensato di soddisfare un mio bisogno di maternità, non ho mai pensato di andare in una clinica in America, di farmi dare un catalogo e di scegliere se il padre di mio figlio doveva essere alto, basso, biondo o moro o quale dovesse essere il suo QI. Non ho mai pensato di contattare una donna, magari casualmente in un momento di difficoltà economica, e di farle affittare il suo utero per impiantare il mio ovulo, mio figlio. Ognuno può vivere la propria sessualità e i propri sentimenti come meglio crede; ma, quando parliamo di azioni che ricadono sulla vita di altri, di scelte che ricadono inevitabilmente sul futuro di neonati e bambini che non possono opporsi, non è accettabile. Noi abbiamo l'obbligo morale di tutelarli anche per il futuro. È immorale approfittare delle difficoltà di una madre per affittare il suo utero per generare un figlio altrui; è una cosa che non sarebbe accettabile nemmeno nel regno animale. E, quando quel bambino chiederà di sua mamma, cosa gli verrà risposto? Tu sei un bimbo speciale: non hai una mamma, ma due papà. Oppure hai due mamme. scusate, bisognerà rispondere, per essere coerenti: hai un genitore 1 e un genitore 2. Meno male che la natura poi si regola e l'adolescenza presenta il conto di queste aberrazioni, che sarà salatissimo sia per i malcapitati figli che per la coppia che li ha voluti. Lo Stato non può prendersi la responsabilità di tutto questo. Io voglio un mondo dove i bambini possano ancora dire mamma e papà, senza sollevare un polverone, e voglio continuare a dire che la natura ha disposto per la specie umana un padre e una madre e che esiste solo questa possibilità biologica. Il resto è una manipolazione egoistica. Io non voglio che nessuno vada a scuola a dire a mio figlio che non è un maschio, ma che deciderà il suo sesso in seguito. Nessuno deve permettersi di invadere la sfera educativa di mio figlio, che è disciplinata da suo padre e da sua madre. State lontani dai bambini. Voglio ricordare che l'onorevole Zan qualche giorno fa ha dichiarato che ci sono bambini e bambine che percepiscono un sesso diverso dal loro sesso biologico e che dobbiamo aiutare questi bambini in un percorso di transizione. Ecco la vera intenzione. Io aiuterei proprio lui a risolvere tali conflitti dentro di sé, visto che è già da tempo in età adulta. La natura fa il suo corso anche per questi dubbi, che esistono e che vanno risolvendosi non occorre l'aiuto di nessuno per fare ciò che la natura ha già disposto. L'unico aiuto che possiamo dare è studiare forme di sostegno psicologico e culturale per i genitori che ancora non rispettino le identità sessuali dei figli, perché il rispetto dell'identità sessuale è un dovere ed è un percorso rivolto eventualmente ai genitori e non ai figli, ai quali pensa già la natura con la sua perfezione. Un figlio nasce dall'amore di un uomo e di una donna che decidono di donare la vita: voglio continuare a dire tutto ciò, senza essere tacciata di omofobia. È doveroso e necessario rispettare dei limiti etici, che non possono essere superati dall'egoismo personale e dal narcisismo e tutto questo non ha nulla a che vedere

ringrazio il collega che è salito fino a qui e mi ha consigliato di non arrabbiarmi, perché seguirò il suo consiglio, che ho apprezzato molto. col piede sbagliato, perché quando si parla delle persone, della loro sofferenza e dell'identità intima di ognuno,

di ciò che è vero e concreto. Qui non si tratta di imporre agli altri la nostra visione del mondo, ma di accettare il mondo per quello che è. Non si tratta di stabilire se le carriere dei magistrati debbano essere o meno divise: questa è una visione politica. In questo cercando di approvare un atto legislativo che, nella sua definizione, sia dissuasivo di azioni di odio verso persone che, non per scelta ma per natura, hanno una percezione diversa della propria sessualità. Stiamo provando, con un disegno di legge, a fare un atto di cultura, per far comprendere a tutti che non siamo tutti tutti binari e che ci sono persone che, non per scelta ma per nascita, per il proprio sentire, una strada di transizione. Questa strada di transizione, naturalmente, porterà ad una definizione e a un'identità diversa rispetto al sesso di nascita, ossia il sesso biologico.

Non è però un neologismo, tanto che in Europa sono già 11 i Paesi che prevedono tutele per l'identità di genere (sono 20, se consideriamo il Consiglio d'Europa). In Europa se ne sta parlando dal 2000 nel 2010 il Comitato dei Ministri fece una raccomandazione per misure legislative di contrasto ai crimini d'odio - questo è il nostro caso - per l'orientamento sessuale e l'identità di genere.

in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». Mi accorgo che molti parlano senza conoscere i fatti. Cosa c'è dietro questa

perché la nostra legge prevede che soltanto all'atto finale della transizione l'identità di genere sia riconosciuta, mettendo queste persone in condizione di non poter accedere al mondo del lavoro. Questo non risolve la questione, ma è un primo passo, in quanto la riconoscibilità della propria identità di genere anche in una frase di transizione non conclusa è un fatto fondamentale. Stiamo compiendo un atto culturale, ci sono persone costrette a vivere nell'illegalità, nella prostituzione, come gli invisibili presenti sul nostro territorio a causa di alcuni decreti

che stanno facendo un percorso di transizione e vengono esclusi dal mondo. Questo è un dato ed è sulla pelle della gente, sulla pelle delle persone, sulla loro sofferenza. È inutile, poi,

questa specifica che è stata introdotta alla Camera per rassicurare quelli che ritenevano che l'opinione sarebbe stata perseguita, che non ci sarebbe più stata

e sempre tutelato, e ci mancherebbe altro! Quello che non si può fare è istigare all'odio e si parla di reato di pericolo concreto. Neanche questa è un'espressione nuova, perché fa parte del nostro ordinamento giuridico, nel quale i reati sono divisi in pericolo astratto, in pericolo concreto e in danno e questo ambiti, anche per il danno ambientale c'è il pericolo concreto e sono fattispecie già presenti nel nostro ordinamento, sono conosciute. Ebbene, se il pericolo viene giudicato astratto, il reato non sussiste, quindi è chiaro che è il giudice che dovrà valutare, perché c'è la divisione dei poteri, la legge non può imporre al giudice come dovrà valutare - vivaddio - ma se il giudice riterrà che non c'è un pericolo concreto, ma che il pericolo di istigazione all'odio è solo astratto, il reato non sussiste e un'opinione non può mai essere un'istigazione all'odio, semmai lo volesse essere. Quanto all'articolo 7, non c'è alcun obbligo per le proposte operative nelle scuole, c'è soltanto una possibilità e questa è l'azione anche più importante della legge, perché oltre ad essere punitiva una legge è dissuasiva, ma soprattutto è un atto culturale, perché noi potremo sconfiggere l'isolamento, la frustrazione e l'odio solo con la conoscenza e la conoscenza la si persegue attraverso la scuola, attraverso operazioni culturali che coinvolgano le persone, i bambini e rendano loro nota la realtà, perché questa non è un'invenzione culturale, non è

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16,30

Per questa votazione ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale indicherà, ai sensi dell'articolo 49, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un solo nominativo tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nell'ambito della procedura di selezione prevista dal comma 6-*bis* del medesimo decreto legislativo, il cui *curriculum* è pubblicato nel sito Internet del Senato. Avverto che, avendo taluni candidati lo stesso cognome, ove si intenda votare per uno di essi occorrerà indicare sulla scheda, ai fini dell'attribuzione del voto, sia il cognome che il nome dell'interessato. In mancanza dell'indicazione del nome il voto sarà considerato nullo. Saranno proclamati eletti i due candidati che otterranno il maggior numero di voti. Dopo la chiama le urne resteranno aperte fino alle ore 19,30, mentre l'Assemblea proseguirà nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno. Dichiaro aperta la votazione e invito il senatore Segretario a procedere all'appello

Messina Assuntela, Mininno,

«La mia libertà finisce dove inizia la vostra». Queste sono le parole di Martin Luther King, un uomo che ha sacrificato la sua vita per combattere le discriminazioni, diventando simbolo della lotta al razzismo e a tutte le forme di discriminazione. Fratelli d'Italia non ha mai posto in discussione la libertà di ognuno di vivere la propria sessualità come meglio crede: non è certo questo il punto della discussione. Ciò che riteniamo inaccettabile è quando si tenta, attraverso lo Stato, di imporre determinati modelli alla società, di cui francamente non si sente il bisogno. La nostra contrarietà nasce dal fatto che questo impianto normativo è giuridicamente sbagliato, in alcuni punti anche incostituzionale e fondato su principi distorti per la tutela delle libertà e su rimedi sbagliati per il contrasto alle discriminazioni. Ci sono alcuni episodi, certamente da condannare - ma non sono prevalenti: sono molto più numerose le violenze sulle donne o sui minori, tanto per fare un confronto - che vengono regolarmente perseguiti, anche aspramente, nell'attuale quadro normativo. Infatti le norme attuali sono perfettamente in grado di colpire già oggi, con maggiore forza, eventuali episodi di violenza di questo tipo, ad esempio inserendo le aggravanti per futili motivi, senza dover inventare una nuova fattispecie. A nostro avviso il disegno di legge Zan è dannoso, perché ideologicamente orientato ad imporre un punto di vista sulla realtà, cancellando posizioni differenti. La totale incertezza giuridica del cosiddetto reato di omofobia rende l'applicazione della legge estremamente incerta affidata all'interpretazione del giudice, esponendo così legittime affermazione di libertà di opinione al rischio di essere tacciate di omofobia. Un ulteriore punto controverso, sul quale poniamo la nostra ferma opposizione, è l'impianto propagandistico e rieducativo di tante parti del testo, che non si limita a chiedere pene più pesanti per atti concreti di violenza, ma costruisce tutta una serie di attività di propaganda *gender,* come la Giornata nazionale del 17 maggio, i corsi nelle scuole anche ai bambini di dieci o dodici anni e la rieducazione di chi viene condannato. Basta leggere una sola volta questo testo, per capire il carattere controverso del principio sotteso. sotteso. Perplessità sorgono anche per la parte in cui si dice «ai fini della presente legge», perché ciò costituisce un'oggettiva limitazione alle frasi che seguono, che sono invece diritti costituzionali irrinunciabili. Se le opinioni espresse non sono ai fini della legge in questione, questa libertà decade? Ma chi decide in questa corrispondenza, visto che la legge è costruita su concetti giuridicamente sdrucciolevoli come l'omofobia, la cui definizione, tra l'altro, il nostro ordinamento ancora non ha concepito o, come riportato all'articolo 2, sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, concetti anch'essi ancora non definiti giuridicamente e sui quali non c'è ancora convergenza nemmeno all'interno della stessa comunità LGBT. La società via via si adeguerà, con la gravosa conseguenza che non esisteranno più i membri di una Nazione che sono uguali davanti alla legge nazionale e si riconoscono in una storia comune, per poi riconoscere altrove una umanità comune che è radice feconda delle proprie differenze. Assisteremo ad una polverizzazione della società in una miriade di sottoinsiemi che non si incontreranno e non si troveranno, che egoisticamente e narcisisticamente guarderanno solo a sé e alla propria autoaffermazione, pretendendo unilaterali riconoscimenti e distruggendo la trama del legame sociale che la storia pazientemente si era occupata di tessere. Ecco allora che ciascuno dipinge sulle sue mani il nome di una giustizia di parte che cede alle lusinghe della difesa di vittime che vittime non sono più. Di fronte a ciò e di fronte a un progetto di legge evidentemente sbagliato, che distingue i reati non in base alla qualità dell'azione, presupponendo che si debba sempre tutelare il valore unico della persona, ma in base alla categoria di appartenenza della vittima, non si deve transigere. Più si legge il testo, più emerge il carattere ideologico di questa legge, in quanto tale sarà potenzialmente dannosa sia dal punto di vista culturale che sociale. In primo luogo, pensare di introdurre in tutte le scuole iniziative contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia nella giornata nazionale fissata ogni anno il 17 maggio significa far entrare nei percorsi scolastici anche delle classi elementari e medie contenuti in linea con l'impianto della legge, che sono tutt'altro che universalmente condivisi, come succede invece per le giornate contro la mafia e l'antisemitismo, arrecando quindi una dubbia comprensibilità da parte dei bambini, ai quali si finirebbe per far credere che le esperienze che vanno facendo della realtà sono una finzione, essendo l'umanità non declinata al maschile e femminile ma oggetto di infinite identità, tutto questo in un'età nella quale si va formando la percezione di sé in relazione a ciò che li circonda. È ovvio che nelle intenzioni del proponente si è reso indispensabile farlo perché troppo troppo vaghi erano i concetti sui quali si intendeva costruire niente meno che fattispecie penali, con la pretesa di educare a colpi di codice. Il problema allora sta proprio in questa intenzione di perseguire come discriminatorie quelle che di fatto sono concezioni differenti della natura umana, oggetto di legittimo confronto e di convinzioni profondamente radicate nella coscienza di tanti cittadini. Qui come in un precipizio di estrazioni ideologiche connesse le une alle altre entriamo fatalmente nel campo della libertà di opinione, sulla quale si è tentato si è tentato di apporre lo scudo protettivo in una sorta di salvacondotto, che però non basta. Troppo largo, infatti, è lo spazio per l'interpretazione discrezionale discrezionale di cosa possa istigare ad atti discriminatori o persino alla violenza. Numerose sono le domande che ci stiamo ponendo sulle conseguenze di tale normativa: chi stabilisce dove e come si può esercitare un dissenso rispetto a quella che diviene una legge dello Stato? La scuola paritaria che non vuole celebrare la giornata anti-omofobia può farlo o è destinata a pagare una sua intangibile libertà? Sarà ancora lecito per un sacerdote esprimere nella predicazione, a un catechista nella sua classe, a un insegnante a lezione, a un genitore con i propri figli concetti che potrebbero essere tacciati di omofobia? La femminista che oggi contesta alla radice il concetto di identità di genere potrà ancora farlo pubblicamente? Ciò che rende insopportabile l'impianto di questa legge è la palese violazione di un diritto costituzionalmente garantito come la libertà del proprio pensiero, così come cristallizzato dall'articolo 21 della Costituzione. Infatti, l'aspetto più problematico del disegno di legge Zan è che il pensiero unico prodotto dal politicamente corretto vorrebbe limitare ogni dibattito. In poche parole, chiunque esprime un parere diverso da quello dei promotori della legge viene immediatamente tacciato di omofobia e le sue ragioni sminuite o escluse dal dibattito pubblico. Concludendo, noi di Fratelli d'Italia diciamo di no alla proposta del disegno di legge Zan perché mette in discussione in modo pericoloso l'espressione della libertà di pensiero garantita dall'articolo 21 della Costituzione.

il disegno di legge Zan in approvazione in questa Camera rientra a pieno titolo nella cultura tipica della sinistra che punta a cancellare l'identità e a punire e perseguitare chi non la pensa allo stesso modo. Da mesi la sinistra prova a imporre il pensiero unico e, se non la pensi allo stesso modo, sei tacciato di razzismo, omofobia, transfobia e chi più ne ha più ne metta. Il guaio di questa sinistra è che in ciò che fa è subdola e questo testo ne è un esempio lampante. Il disegno di legge Zan nasce con tutte le buone intenzioni di difendere delle persone che si sentono discriminate, ma finisce per condannare tutto il resto del mondo. Che sia una legge che fa tutt'altro rispetto al condannare le discriminazioni lo si evince chiaramente dall'articolo 1 che ha la pretesa di essere meglio di Wikipedia, definendo cosa sono il sesso, il genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Veramente voi avete la pretesa di racchiudere concetti così vasti in un articolo e renderli norma di legge? Forse serve ricordarvi che abbiamo in Costituzione un articolo che disciplina le uguaglianze. Lo fa senz'altro meglio. Serve davvero il vostro articolo 1 di questo disegno di legge? È ancora peggio l'articolo 4 del presente disegno di legge. Dite che sono fatte salve la libera espressione di convincimento od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. E meno male. Poi aggiungete che tutte le idee e le opinioni vanno bene, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. diciamo chi stabilisce cos'è un concreto pericolo. Quando è che un pensiero può incitare un atto violento? Quali sono i parametri di riferimento? La vaghezza di questo articolo crea un vuoto che è una seria minaccia alla libertà di espressione. Siete riusciti a calpestare persino l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero e ciò che è peggio è che lo avete fatto in nome della difesa di soggetti che considerate deboli e che, invece, state usando come scudi umani. Al contrario di ciò che qualcuno vuole far credere, noi non siamo omofobi, transofobi o razzisti, noi siamo per il rispetto delle idee e voi il rispetto per le idee lo cancellate. Noi siamo per la libertà: amate chi volete, fate ciò che volete del vostro corpo; a noi interessa poco, ma possiamo essere liberi di dire che la famiglia è fondata sull'unione di un uomo e di una donna? Possiamo essere liberi dire che la pratica dell'utero in affitto è una barbarie? Possiamo dire che è un'ingiustizia che un atleta, nato biologicamente uomo, competa con le donne solo perché si sente donna, falsando quindi l'esito delle gare? Possiamo essere fieri di essere mamma e papà, invece di nasconderci dietro «genitore 1» e «genitore 2»? Possiamo sostenere tutto questo o dobbiamo chiedervi il permesso? Possiamo esprimere le nostre opinioni senza temere che un giudice ci accusi di istigare odio? Ecco, noi rivendichiamo il diritto di ciascuno ad amare come crede, a chiedere rispetto del proprio amore, ma questo non significa aver timore di sostenere le proprie idee. Per noi la libertà di amare è sacra, come è sacra la famiglia, come sono sacri i bambini. Non facciamo gerarchie, ma investiamo sul futuro e vogliamo lasciare ai nostri figli la possibilità di costruirsi il proprio futuro senza che noi glielo imponiamo con le ideologie di oggi. Voi invece avete la pretesa di sottrarre l'educazione ai genitori per istituire nelle scuole una giornata dedicata all'ideologia *gender*; le stesse scuole dove non si insegna educazione sessuale. Siate seri, lasciate fuori i più piccoli da questa norma di legge, anche perché le ingiustizie non si cancellano mai con delle iniquità: la legge deve avere misura e chi va contro la legge che evidenzia prepotenze deve essere punito e basta. A dirla tutta, la legge vigente già prevede punizioni per chi discrimina, per chi offende, per chi usa violenza, a prescindere da chi sia il soggetto che ha subito quelle violenze. Signor Presidente, le leggi per noi ci sono già. Volete migliorarle? Invece abbiamo davanti un disegno di legge che non farà che alimentare polemiche e storture. Noi oggi siamo chiamati a varare una norma contro la violenza e proprio per questo dobbiamo essere rigorosi nel non crearne di nuove, di violenze. Ma voi purtroppo questo vi ostinate a non capirlo. Che poi, a ben vedere questo disegno di legge non piace neppure a voi che l'avete fatto. Siete talmente confusi che non sapete più se il vostro *leader* è Enrico Letta, Matteo Renzi o Federico Lucia, in arte Fedez. Vi fate dettare la linea politica dagli *influencer*,

La verità è che la sola forza di opposizione in questo Parlamento è Fratelli d'Italia, mentre voi dovreste avere i numeri schiaccianti per approvare questa legge; ma così non è e lo abbiamo visto in queste ore. Se siamo arrivati fino ad oggi è perché, quando dicevamo che questa maggioranza era troppo diversa per stare insieme, avevamo ragione e il disegno di legge Zan non è che l'ennesima prova di tutto ciò. Siete una maggioranza che sta insieme per evitare il voto, che non ha idee e quelle poche che ha sono pure confuse, contorte e pericolose, come dimostra questo testo di legge che è in approvazione. quanta ipocrisia in questi banchi. Gli stessi che oggi si ergono a paladini, a difensori dei diritti degli omosessuali, che condannano Orbán per aver fatto una legge contro la diffusione della propaganda LGBT e condannano Giorgia Meloni che coerentemente non rinnega il legame con Orbán, non si stracciano le vesti quando si tratta di fare accordi con Paesi come il Qatar, dove giocheremo i prossimi mondiali di calcio, o l'Arabia Saudita, dove - badate bene - non solo l'omosessualità è un reato, ma è anche punita con la morte. Anche su questo voi chiacchierate mentre noi facciamo i fatti.

gli Stati che prevedono nei loro ordinamenti il reato di omosessualità e non stringa con loro accordi di cooperazione culturale. Vediamo se avremo il supporto unanime di tutti coloro i quali oggi si sentono paladini dei diritti LGBT. Una comunità la si difende sempre e non a corrente alternata. Signor Presidente, davvero si può pensare che questo disegno di legge Zan combatta la discriminazione? Questa norma è un tentativo di indottrinare le persone a pensare in un certo modo, cancellando le loro identità, le culture, le conquiste, per rendere tutti noi nient'altro che numeri e codici. Noi a questa vostra deriva non ci stiamo e non ci staremo e ci batteremo con tutte le nostre forze per impedirla. *(Applausi)*. di legge Zan, questo sconosciuto, credo sia stato l'argomento più dibattuto ultimamente in TV e in ogni dove, ma pochi, pochissimi si sono presi la briga di leggerlo. Voglio portare all'attenzione di quest'Assemblea un aspetto che al momento nessuno ancora ha sottolineato: che ricadute avrà sul mondo imprenditoriale? Più si analizza nel dettaglio il e più insidie nascoste emergono. Ce n'è per tutti, anche per le partite IVA, ovvero i lavoratori autonomi del mondo dell'impresa, della professione, dell'artigianato, del commercio e via elencando. L'articolo 8 prevede espressamente che l'ente governativo denominato ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, noto come UNAR, elabori con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro e alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. Per capire di cosa si tratti in concreto, basta considerare che nel 2013 lo stesso UNAR ha già elaborato una strategia nazionale proprio nei quattro ambiti indicati dal disegno di legge Zan che sono stati definiti assi: educazione e istruzione, lavoro, sicurezza e carcere, comunicazione e media. Vediamo quindi cosa prevede il secondo asse di quella strategia cui il disegno di legge Zan vorrebbe dare valore legale tramite l'articolo 8, ossia quello del lavoro privato, costituito da piccoli, medi e grandi imprenditori, da professionisti, artigiani, commercianti e partite IVA in generale. Il documento dell'UNAR pone l'accento sull'importanza delle pratiche di *diversity management*, favorisce l'attivazione dei talenti e incrementa la produttività aziendale sul cosiddetto *business* inclusivo. Seguiranno sicuramente corsi di informazione per sensibilizzare i datori di lavoro, le figure dirigenziali, i lavoratori e le lavoratrici e le associazioni di categoria sulle tematiche LGBT, nonché la creazione di *network* LGBT all'interno delle aziende e l'istituzione a livello di alta dirigenza del ruolo di mentore LGBT. Non potrà mancare poi la solita opera rieducatrice e allora ecco corsi di sensibilizzazione e formazione per i dipendenti e per tutti i livelli di *management* che aiutano a costruire programmi di *mentoring* e a migliorare i propri percorsi professionali; iniziative specifiche di formazione professionale per transessuali e *transgender* e pubblicazioni informative rivolte ai datori di lavoro. Si capisce molto bene come dietro questa strategia si nasconda, in maniera neanche troppo velata, il *business* dei consulenti aziendali, dei formatori professionali, dei certificatori di tutta quella pletora di soggetti disposti, previo profumato compenso, a spiegare come imprenditori e professionisti dovranno mettersi in regola con le disposizioni dettate dall'UNAR, un po' come quello che è successo in passato con la legge n. 626 sulla sicurezza sul lavoro e con la normativa sulla *privacy*. Ma davvero pensate che imprenditori, professionisti, artigiani, commercianti e lavoratori autonomi di vario tipo non abbiano nulla da dire su questo ulteriore fardello burocratico che verrebbe loro addossato nel caso passasse definitivamente il disegno di legge Zan così la ricaduta sul popolo che vive nel mondo reale poco o nulla interessa al legislatore, preoccupato più che altro di piantare una bandierina ideologica, noncurante di fastidi, costi e incombenze che potrebbe provocare ad aziende, soprattutto medio-piccole, già provate dalla pandemia. Resta sempre più chiaro, dal mio punto di vista, il vero obiettivo di questa proposta di legge che non ha nulla a che vedere con la tutela penale di omosessuali e transessuali. Tre sono le vere ragioni del disegno di legge Zan: indottrinare non solo la scuola ma l'intera società; imbavagliare chi osa dissentire rispetto al pensiero unico *gay friendly*; mettere in piedi un *business* milionario. Insomma tre ottime ragioni, queste, per dire no a questo sciagurato e liberticida disegno di legge.

il tema dell'omofobia è molto serio, come tutte le forme di discriminazione, ma nella fattispecie non si riesce purtroppo a discutere in modo sereno le problematiche sollevate da questo disegno di legge perché, in fondo, il fine non è tutelare le persone dalle discriminazioni, ma imporre posizioni ideologiche su materie che c'entrano poco o niente con l'omofobia. Il problema del disegno di legge Zan è che non è un provvedimento contro la violenza e contro la discriminazione nei confronti degli omosessuali - tema su cui occorre essere molto sensibili e attenti - ma è un disegno di legge

è accaduto anche che un papà abbia trascorso una notte in carcere perché indossava una maglietta con sopra stampata un'immagine di famiglia tradizionale. Quindi il vero tema è stabilire quale sia il vero confine tra discriminazione e legittima libertà di opinione, limite che in questo disegno di legge, a nostro parere, non si pone proprio nell'impedire ogni libertà di espressione su temi per noi fondamentali. Fratelli d'Italia vuole combattere la violenza e la discriminazione, e per questo ci siamo, tant'è vero che abbiamo presentato anche una mozione per condannare tutti quei Paesi dove ancora l'omosessualità è considerata un reato, a volte punita con l'ergastolo e a volte addirittura con la morte. Ma su questo piano non abbiamo trovato una sinistra così sensibile. La sinistra, invece, continua insieme alle associazioni LGBT a denunciare un aumento di discriminazioni e crimini omofobi, smentiti invece dai dati; e non dice una parola, una che sia una, sul mondo islamico *(Applausi)*, dove l'omosessualità è considerata un reato a volte punito, come dicevo, con la morte. Questo ci lascia, da una parte, basiti ma, dall'altra parte, dimostra la posizione ideologica di facciata di questa sinistra. Ne prendiamo atto insieme alla stragrande maggioranza degli italiani, che in questo momento ha ben altro a cui pensare. Torniamo al tema. Signor Presidente, vogliamo ribadire la nostra posizione politica su alcuni punti fondamentali: noi non siamo d'accordo sull'attacco alla famiglia tradizionale, come non siamo d'accordo sull'adozione da parte di coppie omosessuali. Non accettiamo questa discriminazione nei confronti della famiglia naturale, perché riteniamo che proprio la famiglia naturale sia la base del nostro sistema sociale su cui si fonda la nostra comunità. Si rischia che, per difendere i diritti di alcuni, si ledano i diritti di molti; in ogni caso, sarebbe un errore. Siamo inoltre contrari alle adozioni da parte di coppie omosessuali, e non lo diciamo perché siamo omofobi, ma perché sosteniamo che i bambini non debbano essere comprati tramite adozioni dai lunghi e costosi *iter* - che tutti ormai conosciamo - tramite l'affitto dell'utero di una donna: questo proprio non lo possiamo accettare. E lo diciamo perché siamo fortemente convinti che un bambino debba avere il diritto di avere un padre e una madre e che questo diritto non possa essere sacrificato al capriccio di adulti liberi di vivere la propria sessualità come meglio credono. Come dicevo, questo tipo di adozioni come conseguenza porta purtroppo alla prassi dell'utero in affitto: questo è inaccettabile perché significa mercificare il corpo di una donna. Tutto ciò non sta bene nemmeno alle femministe di sinistra, che non accettano neppure loro il disegno come sostiene in un'intervista sul «Corriere della Sera» la storica attivista femminista Marina Terragni, la quale ha dei forti dubbi sull'identità di genere e sul *self-id*, che è una sorta di autocertificazione di genere. Presidente, vorrei introdurre anche questo argomento: l'autodefinizione di genere. Colleghi, per caso avete sentito parlare dei 270 detenuti che si dichiarano donne e chiedono di andare nel carcere femminile? Questo è davvero accaduto in California, dove il *self-id* è legge, di legge Zan verrà approvato, potrà accadere anche da noi. Senza parlare, poi, di quei settori - penso allo sport, alle competizioni sportive - giustamente suddivisi fra competizioni femminili e maschili, che non possono essere messe sullo stesso piano agonistico, dove a quel punto, sì, si creerebbero situazioni imbarazzanti, dove la discriminazione andrebbe al contrario a penalizzare le donne nel competere con persone fisicamente maschili. Forse la sinistra non si rende conto delle conseguenze che potremmo avere in molti settori, però - mi sia consentita la battuta - potrebbe essere un modo per risolvere la questione legata alle quote rosa alle elezioni! Ma andiamo oltre, Presidente. Per ciò che riguarda il gender nelle scuole, mi chiedo perché, nella stessa scuola dove si è deciso di non fare l'educazione sessuale, adesso si voglia spiegare cos'è l'omosessualità. Ricordo a me stesso e ai colleghi che i genitori hanno la patria potestà sui figli e ritengo per questo più che opportuno che l'educazione sessuale non debba essere fatta nelle scuole. I bambini che frequentano le scuole primarie

Se passa la legge Zan, si insegneranno a questi bambini le teorie gender, confondendo le menti di bambini in età evolutiva. l'ideologia della sinistra nostrana si scaglia contro la legge Orbán, definendola una legge contro la propaganda LGBT. In realtà, seppur con toni a volte anche duri, è una legge che vuole difendere proprio quel principio di cui parlavo prima: il diritto dei genitori - e non dello Stato - di insegnare ai propri figli l'educazione sessuale. Vi scagliate contro la legge ungherese e non dite una parola contro tutti quegli Stati islamici che concretamente e cruentemente perseguitano gli omosessuali. Un'ultima cosa, Presidente, e mi rivolgo a voi, colleghi senatori, così sensibili al disegno di In questo testo si menziona la disabilità. Nel corso dell'esame alla Camera il disegno di legge Zan è stato integrato con il riferimento alla disabilità. Ti tratta, tuttavia, a mio parere, di un inserimento che appare forzato, anche in ragione del fatto che non viene riportato in alcuni articoli. All'articolo 1, relativo alle definizioni, non si parla delle disabilità; eppure, questo termine andrebbe eventualmente chiarito. Si tratta di una mera dimenticanza oppure certamente no, come ritengo, visto che durante i lavori parlamentari è stato fatto notare anche il mancato richiamo? Vorrei che i colleghi senatori che sostengono di votare a favore dell'approvazione del disegno di legge Zan così com'è spiegassero cosa c'entra la disabilità con l'identità di genere. Spiegatemi voi perché io ci vedo solo un voler mettere il velo davanti agli occhi degli italiani utilizzando i diversamente abili per gli scopi ideologici della sinistra. Torno a ribadire che siamo contrari all'utero in affitto e alle adozioni per gli omosessuali e chiedo a lei, Presidente, se questa è una discriminazione oppure una legittima opinione. proposta Zan diventa legge, non avremo più la possibilità di esprimere il nostro pensiero liberamente perché verrà meno un diritto costituzionalmente garantito, cioè quello della libertà di opinione e di espressione, sotto la minaccia di omofobia. Fratelli d'Italia sostiene che si debbano combattere le discriminazioni di qualsiasi natura, ma protegge convintamente il diritto di un bambino di avere una madre e un padre e crede che l'utero in affitto sia una barbarie. Non vogliamo bavagli,

oggi è bene essere estremamente chiari dopo che molto è già stato scritto e detto, talvolta anche a sproposito, sul disegno di legge Zan. Questo provvedimento, così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati, non è solo inutile, ma risulta anche dannoso perché strumento ideologico e demagogico. In primo luogo, l'Italia non è affatto un Paese ostile alle persone omosessuali, né secondo le graduatorie europee dei Paesi *gay friendly* né, tantomeno, alla lettura dei dati relativi agli episodi di aggressione a persone omosessuali. I dati degli osservatori sono molto chiari in merito; ci sono alcuni episodi, certamente da condannare, ma non sono certo prevalenti. Sono molto più numerose le violenze sulle donne o sui minori, tanto per fare un confronto, che vengono regolarmente perseguite anche aspramente nell'attuale quadro normativo. Le norme attuali sono perfettamente in grado di colpire già oggi con maggior forza eventuali episodi di violenza di questo tipo, senza dover inventare una nuova fattispecie. disegno di legge Zan è dannoso perché ideologicamente orientato ad imporre un punto di vista sulla realtà, cancellando posizioni differenti. La totale incertezza giuridica del cosiddetto reato di omofobia rende l'applicazione della legge estremamente incerta, affidata all'interpretazione del giudice, esponendo così legittime affermazioni di libertà di opinione al rischio di essere tacciate di omofobia. Se affermo che un bambino ha diritto ad un papà e ad una mamma, mi chiedo se sono omofobo oppure no. Se sostengo che non è legittimo reperire all'estero un figlio partorito su commessa da una donna, sono omofobo?

propagandistico e rieducativo di tante parti del testo che non si limita a chiedere pene più pesanti per atti concreti di violenza, ma costruisce tutta una serie di attività di propaganda *gender* - la giornata nazionale del 17 maggio, i corsi nelle scuole anche a bambini di che evidentemente servono a condizionare le libertà di opinioni più che a proteggere le eventuali vittime. Un ultimo punto per cui il disegno di legge Zan va respinto nell'attuale stesura sta nella formulazione del cruciale articolo 3 che, nella versione emendata, recita testuali parole: «ai sensi della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alle libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». In primo luogo dovrebbe allarmare ogni cittadino il fatto stesso di dover scrivere in una legge che è fatta salva la libera espressione. *(Applausi)*. Ci mancherebbe altro in uno Stato democratico e di diritto, per chi crede, come noi, che le libertà dei cittadini siano sancite dalla Costituzione e non da una concessione della politica o di una legge qualsiasi ben più effimera del dettato costituzionale. Per concludere esorto tutti i senatori presenti ad avere un sussulto di orgoglio e di responsabilità personale per negare l'approvazione del testo testo emendato dalla Camera dei deputati, che è sicuramente perfettibile. Si tratta di un provvedimento altamente divisivo soprattutto nel Paese, prima ancora che tra i partiti, e quanto mai inopportuno di fronte alle costanti richieste di responsabilità e di unità nazionale. Qui non si tratta di negare i diritti e tutela a persone quando ne hanno bisogno, si tratta invece di rifiutare una legge che rischia di diventare un tribunale ideologico liberticida senza alcuna reale tutela nei confronti delle persone omosessuali.

di Fratelli d'Italia. Ci tengo anche a dire che sono molte le voci fuori di quest'Aula contro gli esiti illiberali del disegno di legge Zan. Non siamo quindi solo noi. C'è l'appello di oltre 70 associazioni coordinate da «*Polis Pro persona*»; c'è «Lettera150», un *think-tank* di oltre 300 docenti. Ci sono inoltre insigni costituzionalisti e giuristi, che si sono espressi nei mesi e nei giorni scorsi, sostenendo che il disegno di legge Zan cristallizza in norme giuridiche alcune definizioni non chiare ed ancora oggetto del dibattito sul piano scientifico. Il disegno di legge Zan, infatti, rende punibile qualsiasi forma di critica o dissenso rispetto ai temi del provvedimento. Ci tengo a sottolineare ai pochi presenti in Aula che non si parla di aumentare i diritti e le libertà delle persone, ma solo di reati. Vorrei che questo, almeno fuori di qui, fosse chiaro: non si parla di diritti, ma di reati, perché tutto è stato posto sul piano penale e si arriva per questo al paradosso che alcune libertà costituzionali possono essere oggetto di sanzione penale. Gli articoli più pericolosi, più critici, per noi sono sicuramente gli articoli 1, 2, 4 e 7, ma ciò non esclude gli altri; non li potrò trattare tutti, ma qualcosa intendo dirla, in particolare sull'articolo 4, sull'articolo 4, che reca la clausola che ribadisce la punibilità delle opinioni che integrerebbero il concreto pericolo che si compiano discriminazioni e violenze. decidere cosa incita alla violenza e cosa non lo fa rimane una prerogativa del magistrato, il che mi sembra pericoloso. Si lascia quindi ai giudici un ampio potere discrezionale nella valutazione di ciò che è da punire

Se è più facile individuare una discriminazione basata sulla razza o sulla religione, cioè sull'orientamento religioso, è molto più difficile individuare una discriminazione basata sul sesso; infatti non è un caso che la risoluzione ONU del 1966 non aggiunge il sesso accanto alla razza e alla religione, ma l'Italia ha colmato questo vuoto nel momento in cui ha provveduto con la modifica dell'articolo 3 della Costituzione, che però sembra che gli estensori del disegno di legge Zan non riconoscano.

è necessario che la legge descriva puntualmente la condotta illecita e proibita. Non può essere il giudice a definire l'azione vietata e a indicarne gli elementi di fatto. Un giudice può (e deve) valutare la liceità di una condotta, ma non può valutare la liceità di un'idea, a meno che non decidiamo che esiste il reato di opinione, che è quello che gli estensori della legge infatti hanno deciso Un altro punto estremamente controverso, che però mi è particolarmente caro perché lo studio da tempo, è quello contenuto nell'articolo 1. È incredibile che all'interno di una legge si voglia definire cosa si debba intendere per sesso (biologico o anagrafico), per genere (manifestazione esteriore), orientamento sessuale (attrazione per), identità di genere (identificazione percepita di sé). è la seguente: mentre voi elaborate questo articolo 1, qual è il modello antropologico a cui vi richiamate? Praticamente, infatti, il Parlamento sta decidendo e imponendo un modello antropologico, etico e filosofico con queste paroline, quando nessuno di noi per esempio ha pensato mai di imporre un modello antropologico di origini cristiane, nel quale personalmente io credo, ma stiamo, stavamo e vivevamo laico *(Applausi)*. Nel disegno di legge Zan l'identità di genere è soggettiva - lo sottolineo -, si identifica con la percezione che si ha del proprio sesso; dato reale oggettivo è quindi cancellato e si approda, di conseguenza, a un'indifferenza sessuale. Ma non è tutto, c'è di più: la nozione di identità di genere, introdotta dall'articolo 1, è labile, appunto una percezione soggettiva, mutevole e transitoria e tutto può essere percepito come discriminazione rispetto a una nozione così labile e fluida. Questo concetto ricorre anche nelle altre norme del disegno e crea confusione, perché l'unità e l'identità del singolo vengono scomposte in una pluralità di categorie biologiche o naturalistiche, dimenticando per esempio una cosa: la tutela costituzionale della persona.

il gioco è molto chiaro, ma va un attimo rovesciata questa trappoletta e non c'entra niente l'omofobia; se uno non condivide questo impianto non è omofobo. Qui c'entra il fatto che state imponendo un modello antropologico di un certo tipo; qui c'entra il fatto che nelle scuole, dove non si fa educazione sessuale, si farà l'educazione di genere; qui c'entra il fatto che siamo di fronte alla più grande offensiva ideologica da parte, appunto, dei sacerdoti del *gender*.

un furore così non lo ricordo. Un oltranzismo *gender* che si lega, tra l'altro, alla tirannia del pensiero unico, all'esasperazione del cosiddetto maledetto - aggiungerei - «politicamente corretto»: c'è questo nell'operazione Zan. Zan. È questo il nodo, è questo il punto; il resto è quello che raccontate, è uno *storytelling*, perché qui c'è la volontà precisa di di rieducare, anzi voglio dire di riprogrammare culturalmente i bambini, i giovani, le persone e quindi la società. Quindi, non è in gioco, come raccontate, la libertà di amarsi; non è questo il punto, perché noi non siamo contro questa libertà di amarsi. Qui c'è in gioco ben altro: c'è in gioco tutto quanto sto dicendo e quello che voi chiamate aiuto, che in realtà è una spinta ai bambini a transitare da un sesso ad un altro in in base alla percezione di sé, come se tutti i bambini soffrissero di disforia di genere. Allora è molto pericoloso quello che volete fare, è veramente oltre, perché poi l'orizzonte è chiaro: ideologia *gender* e ditelo, anche se non c'è scritto, che scritto, che poi c'è la missione della maternità surrogata, dell'utero in affitto, dell'adozione delle coppie *gay*. *(Applausi)*. Ditelo che in Europa vogliono inserire questo reato nei crimini d'odio.

nuovi sacerdoti di una società *genderfluid*, in cui nell'indistinto tutto è possibile, tutto è consentito, tranne che pensare e pensare diversamente da quello che voi scrivete. Fratelli d'Italia si batterà ovunque contro questo disegno di legge liberticida, pericoloso e inutile.

ore, anche se mi auguro sinceramente che alcuni colleghi intervenuti siano in cattiva fede, piuttosto che pensare che credano davvero a ciò che dicono. Mi fa paura immaginare che oggi nel Parlamento italiano, nel Senato della Repubblica, si argomenti davvero con questo tipo di argomentazioni una contrarietà che è più che legittima a un provvedimento di legge (ci mancherebbe altro). Ma, per argomentare contro, non bisogna andare a istigare paure e a raccontare chissà quali complotti e ideologie che sarebbero in atto. Qui è tutto molto semplice: su alcune questioni abbiamo delle opinioni diverse, anche rispetto a chi un giorno tende la mano, però poi dovrebbe ascoltare gli interventi dei propri parlamentari, perché io di mani tese oggi non ne ho viste tante e, se erano tese, rischiavano di arrivare da qualche altra parte e non a stringersi. Chi tende la mano propone di limitare l'intervento all'ambito punitivo. Ecco, questo è un punto di differenza: noi pensiamo che la componente educativa e la componente culturale di questo provvedimento di legge siano molto importanti. Quindi abbiamo cercato, con grandissima tranquillità, ascoltando tutti, confrontandoci, cercando di trovare punti di contatto e investendo molto tempo (perché questo provvedimento non lo stiamo facendo con uno schiocco di dita), e abbiamo creduto abbiamo creduto che il Parlamento italiano fosse in grado, nel 2021, di approvare una legge che prevedesse anche la possibilità di aiutare questo Paese a prendere atto che esistono tante forme diverse di stare insieme, di concepire la propria vita, di realizzare il proprio sé, di amare di costruire una famiglia. Tante forme diverse: nella modernità c'è anche questo. Devo dire che negli interventi di queste ore ho sentito tanta paura della complessità, tanto bisogno di ordine, tanto bisogno di oggettività. Però l'ordine e l'oggettività, su cui la filosofia del Novecento ha scritto centinaia di pagine, non esistono più; bisogna prendere atto che esiste il disordine, che esiste il caos, che esiste la complessità e che dentro a questo panorama bisogna vivere con serenità, dando a ognuno la possibilità di trovare la propria strada, senza far credere a nessuno che esistano delle strade giuste e delle strade sbagliate. In questi anni in Parlamento non ho praticamente mai letto. Oggi voglio fare un'eccezione, perché non sapevo che sarebbe successo, ma lunedì ho ricevuto una lettera che mi ha veramente molto commosso. È una lettera che parla di bambini (tanti hanno parlato di bambini in quest'Aula); è una lettera che parla di bambini, scritta da un ragazzo del mio territorio che bambino non è più, ma che si ricorda quando era bambino e quando, da bambino, cercava di capire se poteva essere come sentiva di essere e pensava purtroppo di non poterlo fare. Ve ne leggo solo un pezzettino. Questa lettera dice così: «Se a me qualcuno a scuola mi avesse detto che anche noi possiamo esistere come gli altri, che anche noi siamo una valida possibilità nel mondo e nella società, la mia vita avrebbe avuto molte meno sofferenze. Ho passato venticinque anni nel segreto e nella vergogna, nell'esclusione, nella paura di essere rifiutato dalla famiglia, dagli amici e dal mondo. E allora vi prego: pensate ai bambini, insegniamo loro a non odiare e a non odiarsi per via della loro identità di genere o della loro sessualità. Facciamo educazione soprattutto nelle scuole per questo». *(Applausi)*. Questo è un punto su cui probabilmente non siamo d'accordo e non riusciamo a trovare un accordo, perché non è che possiamo trovare un accordo indipendentemente da quale sia l'accordo; questo per noi è un punto fondamentale. Riusciremo ad approvarlo? Noi speriamo di sì e faremo di tutto per farlo. Non riusciremo ad approvarlo? Qualcuno si assumerà questa responsabilità, perché la questione è se queste persone hanno la possibilità di esistere. Io ne conosco tanti e tra l'altro so che il mio è un osservatorio privilegiato. Io penso di avere una persona molto cara che ha una storia importante, culturalmente importante, e che ha aspettato però che suo padre non fosse più in questo mondo per potersi dichiarare apertamente omosessuale, perché ha sempre pensato che non poteva dargli un dolore, il dolore di essere quello che era. Ha aspettato che non ci fosse più: questa è l'Italia degli anni 2000. E questa è una persona colta, una persona fortunata, una persona che sta bene. Quante persone così non hanno neanche gli strumenti culturali per capire cosa sta succedendo? Allora noi ci vogliamo davvero fare carico di queste storie?

che i giudici possano sbagliare. I giudici servono a questo e credo che quello al nostro esame sia un testo che permette, nel nostro sistema giudiziario, che è articolato, complesso, con tre gradi di giudizio, di evitare che qualcuno venga punito per reati che non ha commesso. Ho sentito fare un ragionamento anche sullo stigma. Ma certo, ci mancherebbe! Certo, qualcuno si è scoperto garantista negli ultimi mesi,

ma c'è una bella differenza tra esprimere un'opinione e, con la propria opinione, far sì che qualcuno possa essere ferito, colpito, umiliato e magari maltrattato.

se il Parlamento italiano ogni tanto riuscisse a sviluppare anche un pensiero culturale, a leggere la realtà e a capire come deve aggiornarla. La realtà va aggiornata nel senso che oggi la complessità della definizione dell'identità è molto più complicata, da tutti i punti di vista. È complicato definire la propria nazionalità e quindi nel Paese esistono tante persone che sono italiane da molto tempo, ma non siamo ancora riusciti a riconoscere che ci sono e c'è qualcuno che ha difficoltà a farlo. Esistono poi molte persone che, nel corso della propria vita, hanno magari cambiato la percezione di sé.

sarebbe molto bello. Come Partito Democratico - ma lo condividiamo, per fortuna, con altre forze - pensiamo che esista una antropologia della pluralità, della possibilità di essere cose diverse nel corso della propria vita, della possibilità di sperimentarsi e di provare ad assaggiare momenti diversi della propria vita e che tutto questo non possa essere giudicato e condannato. Vedete colleghi, c'è un tempo per discutere e c'è un tempo per decidere. Abbiamo molto discusso: oggi dobbiamo dire al Paese se è maturo per dire che odiare è reato e che educare alla pluralità è un fatto positivo. Signor Presidente, colleghe e colleghi, gli occhi del Paese sono vigili sui nostri lavori, perché oggi discutiamo di un progetto legislativo che sta a cuore a milioni di italiani. Non possiamo, in coscienza, voltarci dall'altra parte. Le grandi battaglie sui diritti civili, come nel caso del divorzio, dell'aborto e delle unioni civili hanno segnato il percorso democratico del nostro Paese e del suo ordinamento giuridico. Ora ci troviamo di fronte ad un testo che va a modificare gli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale e stabilisce l'estensione dei delitti contro l'uguaglianza, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Il tema del maggiore contrasto alle discriminazioni e alle violenze per motivi sessuali non è nuovo.

ci sarà una valida ragione per questo. Al di là dei tecnicismi della proposta di legge Zan, di cui tanti hanno discusso, ci troviamo di fronte a una situazione di fatto che vede contrapposte le fazioni di chi considera il testo inutile e ambiguo e di chi, al contrario, lo reputa non solo opportuno ma anche indifferibile. Il punto della questione è il seguente: sappiamo che c'è stata già una mediazione alla Camera dei deputati in sede di prima lettura ed è stato previsto l'inserimento nel *corpus* normativo dell'articolo 4 che, al fine di evitare ogni interpretazione intenzionalmente dubbia delle nuove disposizioni, tutela la libera espressione di convincimento o d'opinione, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Ciò che intendo dire è che il compromesso sulla formulazione del testo è stato già trovato in sede parlamentare e che, giunti a tale momento, questo ramo del Parlamento non può permettersi di far tornare tutto al punto di partenza come nel gioco dell'oca, se non intende affossare definitivamente il percorso legislativo di un tema che, a ragione, grande parte del nostro Paese ritiene prioritario. Questo appello è rivolto quindi non alla cosiddetta disciplina di Gruppo - le posizioni sono note da tempo - ma alla coscienza individuale di ogni senatore, perché con l'assunzione di questa funzione istituzionale bisogna essere pienamente consapevoli delle conseguenze relative alle responsabilità delle proprie scelte. Le campagne di informazione e le mobilitazioni di moltissime piazze italiane avvenute negli ultimi tempi dimostrano l'importanza dell'approvazione del disegno di legge Zan fuori dai palazzi delle istituzioni, per costruire una comunità più coesa e inclusiva, dove ogni episodio di istigazione alla violenza e di intolleranza viene represso sul nascere. Chi cerca un appiglio nel pretesto del riferimento al concetto di identità di genere inserito all'interno del dispositivo mente a sé stesso oppure, al contrario, manipola i propri interlocutori per non dichiarare apertamente la propria contrarietà sul disegno di legge perché politicamente inopportuno. L'espressione "identità di genere", infatti, ha già trovato ingresso in un testo normativo italiano con il recepimento della direttiva n. 95 del 2011, avvenuto con il decreto legislativo del 2014 sull'attribuzione della qualifica di rifugiato nell'ordinamento penitenziario e nella giurisprudenza costituzionale. Dunque, se restiamo inerti di fronte al pericoloso aumento delle violenze e dei soprusi per ragioni basate sul sesso, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, che rappresentano ad oggi i tre motivi di discriminazione più spesso richiamati, offriamo facilmente il fianco alle iniziative delle destre e di quella parte del Paese, che è minoritaria ma per nulla silente, che semplificando come sempre fino all'inverosimile il messaggio lanciato all'esterno, tende a minimizzare l'importanza e l'impatto di più forti misure di contrasto contro ogni fenomeno di sopraffazione e intolleranza. Non è più il tempo di tergiversare o attendere, quindi, in quanto c'è chi aspetta da questo Parlamento un segnale importante e di netta condanna verso chi odia e istiga alla violenza, calpestando senza ritegno la dignità umana e la libertà di vivere secondo i propri orientamenti.

A mio avviso no. Tuttavia, la sinistra e alcuni manovratori del pensiero - non voglio nemmeno definirli manipolatori - hanno creato una suggestione con informazioni false, inesatte, regolate sulla rete; sono scesi in campo anche gli *influencer* che non conoscono il diritto penale, non conoscono le leggi vigenti in questo Paese e hanno ingenerato nel Paese un convincimento che si basa sul fatto che chi vuole la legge Zan contrasta le violenze, le aggressioni, gli episodi come ce ne sono stati anche recentemente, e chi invece non vuole la legge Zan è aperto alle aggressioni, alle violenze, alle prepotenze. Questa è la grande menzogna che dobbiamo spazzare via perché non è assolutamente vero. Noi abbiamo già nel nostro ordinamento numerose norme che consentono di punire chi compia qualsiasi atto di violenza. Con le aggravanti, quando ci sono motivazioni futili e abiette, si può punire ancora più severamente chi per ragioni di discriminazione, di pregiudizio sessuale o per omofobia - termine che è stato coniato negli ultimi anni - compie delle violenze. Quindi, non è vero che ci sia un vuoto normativo. Sono bugiardi coloro che lo affermano. Che lo facciano degli strimpellatori di terzo ordine può anche andare, ma che dei legislatori alimentino questa menzogna è inaccettabile. Vedo, talvolta, anche nelle nostre famiglie e nella nostra parte politica la suggestione della menzogna che prevale sulla verità. verità. Bisogna spiegare alla gente che, con le motivazioni futili e abiette, si può punire più severamente chiunque; che ci sono norme del codice penale poste a presidio della sicurezza dei cittadini con punizioni severissime e che, per quanto nessuno debba sottovalutare nemmeno un singolo episodio di violenza, i dati statistici diffusi dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori dimostrano che nell'arco di quasi un decennio gli episodi - io non li voglio sottovalutare - si contano nell'ordine di alcune decine. Non c'è un'emergenza gigantesca che giustifica un decreto e, comunque, anche un solo atto di violenza giustificherebbe l'aggravamento delle norme. Volete l'aggravamento delle norme? Lo abbiamo proposto con il testo di legge presentato da alcuni esponenti del centrodestra. Qualcuno ci deve pure spiegare cosa c'entra con la sanzione aggravata e rafforzata di chi compie per motivi di pregiudizio sessuale degli atti di violenza o di discriminazione tutto il resto della legge. L'articolo 1 del disegno di legge Zan tenta di introdurre una rivoluzione antropologica nel Paese con una norma che è più rilevante di un articolo della Costituzione. Vergognatevi del fatto di avere portato in Aula questo provvedimento senza discuterlo in Commissione. Vergognatevi del tentativo di mettere il bavaglio. Ci potete mettere la mascherina, che dobbiamo indossare per ragioni sanitarie, ma non ci faremo chiudere la bocca perché l'articolo 1 è gravissimo. Muta, infatti, la vita del Paese. La Costituzione non contiene in tutte le sue parti articoli così importanti. Ce ne sono di fondamentali;

di identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver compiuto un percorso di transizione. Ci sono persone che cambiano sesso e queste cose vanno riconosciute e accompagnate. Ma, quando non c'è alcuna trasformazione o alcun cambiamento, l'articolo 1 di questa legge introduce una rivoluzione antropologica pazzesca, che non è accettabile, è incostituzionale e la Presidenza della Repubblica mai potrebbe firmare

con un articolo che è più importante di una norma della Costituzione che la sinistra, le sue *dépendance* e aggregazioni di altra natura vorrebbero approvare senza nemmeno fare una discussione vera e approfondita. In Commissione non c'è stata e la facciamo in Aula. L'articolo 1 è aberrante, inaccettabile e discriminatorio nei confronti dei cittadini di questa Repubblica. È incostituzionale e non c'entra niente con la lotta sacrosanta alla violenza. Va spiegato al Paese. Se si approvasse questa legge così come è, ognuno può dichiarare in qualsiasi momento un'appartenenza di genere e di sesso cambiando anche più volte, perché non lo si può impedire a una persona. Si sono fatte molti esempi sugli atleti e sulle quote rosa. Non voglio dilungarmi su questo, ma dico che non si può ammettere una volontà indiscriminata di cambiare appartenenza di genere al di là di qualsiasi apparenza. L'articolo 4 sul pluralismo delle idee e della libertà delle scelte contiene formule giuridiche che illustri giuristi di ogni orientamento hanno criticato. Si dice all'articolo 4: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni»

Caliendo, la vedo silente nel Paese. Ho visto invece gli effetti della minoranza faziosa e condizionata da una ideologia di sinistra, e sinistra come aggettivo. Io non voglio mettere in mano alla magistratura le opinioni. Le aggressioni le puniamo più severamente, le discriminazioni le mettiamo al bando, ma io credo che l'articolo 4, così com'è, metterebbe le opinioni ai fruitori del "palamarismo", ai procuratori nominati nelle maniere ignobili che abbiamo visto. Mi chiedo come mai si indaghi su Palamara e non su Pignatone, che era il procuratore della Repubblica che, secondo il libro di Sallusti, prendeva i cornetti in casa di Palamara Palamara parlando col presidente di sezione del Consiglio di Stato, che doveva decidere sul ricorso per la nomina del procuratore della Repubblica di Palermo. A quando un'indagine su Pignatone per traffico di influenze? Io non voglio che le mie opinioni vadano in mano ai Pignatone di tutta Italia, che hanno violato la legge. Lo dico in Parlamento perché almeno qui lo posso dire e perché è la verità. *(Applausi)*. Ci sono tante altre cose che non vanno.

Non si fa l'educazione sessuale, ma si fa l'educazione transessuale nelle scuole. Si passa all'educazione transessuale, senza passare per tappe intermedie. Si può discutere sull'educazione sessuale nelle scuole, su come introdurla, sugli strumenti critici. La formazione è affidata anche alle famiglie, che in ultima istanza, di fronte a bambini così piccoli, mantengono una sovranità educativa che non può essere cancellata. A che serve l'articolo 7? Facciamo la giornata contro la violenza; facciamo giustamente delle lezioni nelle scuole contro le discriminazioni, ma una cosa di questa natura, introdotta dall'articolo 7,

discutere delle aggravanti, se servono, ma già ce ne sono, perché non c'è il vuoto legislativo. C'è un senso comune che vuole punire più severamente queste vicende? Benissimo, facciamolo. Ma non si può usare questa legge per cambiare surrettiziamente la condizione e la cultura del Paese, con l'articolo 1 e l'autodichiarazione di genere, l'articolo 4 e i reati di opinione, l'articolo 7 e l'indottrinamento *gender*. Noi abbiamo tutto il diritto di opporci a questo disegno di legge. Si torni, quindi, in Commissione a circoscrivere l'intervento nella lotta più ferma, più severa alla violenza e si eviti di stravolgere la vita e la cultura di questo Paese e perfino il diritto naturale. È questo un testo che non solo il Presidente della Repubblica non potrebbe firmare, ma che qualsiasi persona di buon senso, se gli venisse spiegato come stiamo cercando di fare con questo dibattito, capirebbe che è inaccettabile e quindi da bocciare. *(Applausi)*. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà. più grave crisi economica che sta purtroppo travagliando il nostro Paese abbiamo sommessamente cercato di far notare da mesi a questa maggioranza che siamo nel pieno della peggiore emergenza che l'Italia conosca dal Dopoguerra ad oggi. in questo momento c'è incertezza soprattutto per quanto riguarda il futuro di milioni di persone, di milioni di italiani che aspettano che il Parlamento lavori ventiquattr'ore al giorno per dare risposte alle troppe domande di sopravvivenza sanitaria ed economica. Se oggi in quest'Aula si discute delle misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere e sull'orientamento sessuale, significa che evidentemente una parte della maggioranza non si rende conto che in questo momento siete chiusi all'interno del palazzo a disquisire di questioni ideologiche su leggi manifesto, segnando una distanza abissale con il popolo che vive invece fuori e che vi vorrebbe vedere lavorare e fare qualcosa di diverso. Evidentemente qualcuno vive in una realtà parallela, fatta solo di ideologia, anziché la realtà purtroppo drammatica che vivono le persone normali per strada ogni giorno. Ebbene, avete imposto questa questa agenda, sostenendo - dal mio punto di vista senza motivo, e lo stiamo dicendo ormai da tanto tempo - che vi siano un'emergenza e un vuoto normativo, quando è evidente invece che non è così. Consultando numerose statistiche e segnalazioni, emerge che le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale sono una parte minoritaria rispetto ad altri più frequenti casi di discriminazione, e soprattutto che ciò che più conta è che tali discriminazioni sono comunque coperte già ora dal nostro ordinamento e non c'è alcun vuoto normativo. Abbiamo tentato di dirlo e dimostrarlo più volte. Ci sono tantissime sentenze di sede civile e anche penale da cui si evince che in Italia le discriminazioni sono già adeguatamente sanzionate dal nostro sistema. Evidentemente a voi non interessa neanche l'articolo 3 della Costituzione.

categoria che sia più uguale delle altre, che abbia una tutela aggiuntiva rispetto alle altre. Voi volete una legge manifesto, una legge in cui le vostre ideologie siano codificate in una norma penale che possa punire chi non si riconosce in esse. Le leggi

agganciando ad esempio il reato a una condotta che configurasse un pericolo concreto e un'adesione effettiva, a partire dal passaggio alla Camera. Li avete incomprensibilmente ignorati. Sempre in prima lettura alla Camera abbiamo

Invece avete imposto la procedibilità d'ufficio, anche in assenza di un pericolo concreto e di una persona offesa che quereli. Questo è francamente inspiegabile, o meglio si spiega sempre con la volontà di introdurre un reato di opinione, una norma manifesto ideologica che vada anche al di fuori dei principi dei principi di buon senso del nostro ordinamento penale. Abbiamo chiesto poi di estendere anche le condotte discriminatorie. Veniamo quindi al punto: cosa intendiamo per istigazione all'odio e alla discriminazione degli omosessuali? Possiamo considerare una messa celebrata per pregare contro la programmazione di questa legge un atto di istigazione alla discriminazione? Va ricordato a tal proposito l'inquietante episodio di Lizzano, dove una semplice veglia di preghiera ha scatenato all'esterno dei locali parrocchiali un *flash mob* di contestatori, con i successivi interventi della forza pubblica e anche del sindaco del Comune. Possiamo considerare istigazione all'odio e alla discriminazione una pubblica manifestazione contro il fenomeno, ormai assai diffuso e praticato, dell'utero in affitto e anche altro? Colleghi, di fronte a un così labile e incerto confine tra lecito e illecito, potete ragionevolmente escludere che nessun giudice e nessun perseguirà mai sacerdoti cattolici o di altre confessioni religiose, semplici credenti o movimenti laici che si rendano protagonisti, sulla base delle loro convinzioni religiose, di contestazioni più o meno

normativo posto a presidio del baluardo della libertà di pensiero e anche della libertà di opinione deve rimanere il più ampio, evitando con la massima cura di consentire al giudice qualsiasi discrezionalità interpretativa. Non possiamo rischiare che nel nostro Paese sia lecito bestemmiare il Dio dei cristiani come il Dio dei musulmani, ma sia vietato e punito bestemmiare l'utero in affitto. Allora facciamo anche delle proposte: per sradicare questi odiosi episodi bisogna agire soprattutto nella scuola e nella periferia, attraverso i *media,* e insegnando ai giovani e anche ai meno giovani il valore della tolleranza e del rispetto della diversità. Vale dunque la pena introdurre queste modifiche liberticide che hanno in potenza un effetto devastante sulla libertà di pensiero e di opinione, che è uno dei principi cardine dello Stato liberale?

Grazie in tutte le salse quest'oggi e anche nelle settimane scorse. E succederà così, perché in alcune scuole, dove avremo magari presidi e docenti particolarmente intraprendenti, o nelle procure, dove avremo dei magistrati particolarmente orientati ideologicamente, questo potrà accadere: si potrà la soglia di un reato concreto e si andrà a punire invece una libera espressione di pensiero. Per questo noi voteremo contro, perché non è pensabile che una minoranza ideologizzata metta il bavaglio alla maggioranza degli italiani. Speriamo che il Senato - abbiamo ancora tempo - anche attraverso le discussioni dei prossimi giorni e della prossima settimana e direi anche finalmente in questa Assemblea - ponga rimedio a questa follia ideologica e riporti alla normalità cambiando le norme di questa legge o bocciandola: questo è quello che chiediamo. Sicuramente a voce alta e in tutte le sedi noi cercheremo di portare avanti il nostro convinto

il disegno di legge che finalmente oggi approda per la discussione in Aula è una misura urgente e necessaria per arginare, contrastare, prevenire e punire un diffuso e insopportabile fenomeno di violenza. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un assurdo dibattito fondato su un presupposto che non doveva nemmeno essere preso in considerazione, e cioè la necessità di avere una legge mirata a risolvere la massiccia discriminazione subita da una parte dei cittadini. Sì, perché c'è chi nella politica e nella comunità italiana nega che esistano comportamenti di odio e intolleranza fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Ho difficoltà a credere che ci sia chi non ne abbia contezza. Penso piuttosto che vi siano ragioni ideologiche *(Applausi)* che spingono alcuni a etichettare in modo diverso, sottostimandoli, gli episodi con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Parliamo di autentica violenza fisica e psicologica; atti che possono minare o distruggere la vita, la serenità e l'equilibrio interiore di una persona. Colleghe, colleghi, purtroppo, chi fonda la propria azione politica sulla parola «libertà», termine spesso abusato o utilizzato senza conoscerne appieno il significato, dovrebbe comprendere bene l'obiettivo di questa legge: ogni persona deve avere la libertà di vivere ed esprimere la propria sessualità, la propria essenza. Che questo spesso venga impedito o represso attraverso privazioni, derisioni, pubbliche umiliazioni, ghettizzazione e anche violenze fisiche è un orrore. Le sceneggiate alle quali abbiamo assistito all'interno delle istituzioni rappresentano un fallimento della politica. Il disegno di legge contro l'omotransfobia ha vissuto mesi di tensione e un autentico calvario legislativo in Senato, in particolare nella Commissione giustizia. Chi non è informato potrebbe pensare che si sia trattato di un normale confronto tra diverse posizioni politiche che, al cospetto di una nuova proposta, esprimono il proprio orientamento. Sappiamo bene che, invece, non è stato così. Questo testo è nato alla Camera molto tempo prima. È il frutto di un lungo confronto di merito che ha visto tutte le forze politiche dialogare, anche sulla base del parere ricevuto da importanti giuristi. Sono state confrontate diverse proposte di legge, tra cui quella del MoVimento 5 Stelle. È stata svolta un'istruttoria in punta di diritto, oltre che sociologica. Si è giunti a un testo base che ha superato il percorso in Commissione e in Assemblea senza clamori e senza particolari problemi. I colleghi di Italia Viva sanno molto bene che le proposte che oggi ripropongono erano state superate con il loro stesso consenso in quel percorso fatto alla Camera. Arrivato in Senato, il testo è diventato oggetto di un duro contendere. Perché? A mio avviso, la destra - la Lega in particolare - ha scelto deliberatamente di farne una questione ideologica, cercando consensi nei sottofondi più oscurantisti del Paese. Ma in questo modo dovete assumervi la responsabilità di fronte a persone che soffrono a causa di frustrazioni, dolori, paure e persino ferite sul loro corpo. Presidente, nessuno meglio di noi del MoVimento 5 Stelle sa che la Lega, fin dall'inizio della legislatura, afferma convintamente che il contrasto all'omotransfobia non è affatto una priorità; anzi, c'è chi nega proprio che esista questa forma di intolleranza. Sappiamo infine che quello perpetrato dalla Lega in Commissione giustizia è stato un autentico ostruzionismo per far perdere giorni, settimane e mesi, al solo fine di boicottare il percorso legislativo. Questa è la verità e l'abbiamo visto anche ieri e oggi. La realtà è che, dietro a vuoti proclami, alberga una sottocultura machista e omofoba, che non vuole estendere i diritti a determinate categorie. Come possiamo credere alle parole di Salvini sulla tolleranza e l'uguaglianza dopo che ha firmato quell'osceno documento con il presidente Orbán? Perché avete paura di esprimere fino in fondo in pubblico la vostra ideologia reazionaria anacronistica, della quale in Europa andate tanto fieri? Servirebbero meno ipocrisia e più coraggio anche per idee che di coraggioso non hanno alcunché, ma che quantomeno ci si deve assumere la responsabilità di avere. Permettetemi di invitare coloro che queste idee le hanno ad aprire il loro cuore, ma soprattutto il loro cervello per capire che garantire diritti non significa toglierne a loro e che questa legge, al di là delle falsità che sono state dette, permette tutti di essere tutelati nell'espressione del proprio io, esattamente al pari delle tutele implicite di cui gli eterosessuali godono ogni giorno senza accorgersene. Oggi il senatore Pillon ci ha raccontato tante storie, anche brandendo la sua fede, ma ha furbescamente evitato di citare le parole del Papa. Dice Francesco che gli omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia; a nessuno deve essere negata questa possibilità.

Sgombriamo il campo da insopportabili tatticismi e ritorniamo tutti insieme ad osservare il problema che lì fuori colpisce molti nostri concittadini. Qualche cifra può aiutarci a comprendere meglio: ogni giorno arrivano circa 50 richieste di aiuto da persone colpite da episodi di omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. Sono circa 20.000 casi l'anno; casi che devono diventare reati. Concludo dicendo che per il MoVimento 5 Stelle la scelta da fare in quest'Aula è obbligata. Noi ci schieriamo ancora una volta dalla parte dei diritti che devono essere sempre rafforzati ed estesi. Ogni cittadino ha il sacrosanto diritto di vivere con serenità, senza soggezione o paura, la propria sessualità. È giunto il tempo di liberarci da un'anacronistica sottocultura medievale. Colleghe e colleghi, siamo nel 2021: approviamo il disegno di

Signor Presidente, intervengo brevemente per portare l'attenzione dell'Assemblea su una situazione abbastanza grave che sta avvenendo nel mio territorio, e in particolare negli uffici giudiziari del tribunale di Monza. «Ci vorrebbe un vaccino per la giustizia monzese»: queste sono le parole del presidente dell'ordine degli avvocati di Monza, che alcune settimane fa ha lanciato una lettera aperta per denunciare l'assoluto abbandono degli uffici giudiziari. Ricordo, in particolare, che il tribunale di Monza è il sesto tribunale su 140 per bacino d'utenza e comprende la mia Brianza, la mia terra popolosa e laboriosa, ed è al ventunesimo posto come organico di magistrati. magistrati. Il presidente dell'ordine degli avvocati lamenta - peraltro concordemente anche con il presidente del tribunale e tutti i rappresentanti degli uffici giudiziari - un organico amministrativo di 86 persone operative su 152. I risultati effettivi di questa carenza sono che, per avere anche solo un'udienza di sfratto o di pignoramento presso terzi, devono decorrere oltre otto mesi.

una macchina per correre ha bisogno di benzina e, in particolare, all'interno dei tribunali la benzina sono le persone, le risorse umane che vi lavoravano e che portano avanti il lavoro per la tutela dei cittadini. Ricordiamo che i tribunali non sono altro che il luogo in cui il diritto e la tutela dei cittadini devono trovare forma e piena attuazione. Lancio questo grido d'allarme sentiti tutti gli operatori della giustizia monzese di cui mi faccio portavoce. So che il ministro Cartabia è molto sensibile su questo aspetto, lo è il Sottosegretario oggi qui presente. Lancio comunque questo grido d'allarme perché non possiamo abbandonare tribunali così importanti come il tribunale di Monza, lasciando sostanzialmente la giustizia così come l'aveva lasciata il predecessore del ministro Cartabia che, nonostante i ripetuti appelli e le ripetute richieste, non ha sostanzialmente fatto nulla. Confido che il Ministero possa muoversi e agire affinché questo tipo di carenza venga meno e, quindi, il diritto e la giustizia possano trovare piena attuazione anche sul territorio monzese.

Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, dal primo luglio, a seguito dello sblocco dei licenziamenti, in varie zone d'Italia sta accadendo quello che temevamo: molte aziende stanno chiudendo e le maestranze sono abbandonate a sé stesse. Dopo i casi di GKN e Gianetti, oggi è toccata alla Whirlpool di Napoli. Sulla crisi dello stabilimento napoletano rimbombano ancora gli annunci sui *social* da parte dell'ex Ministro e del suo successore, che garantivano soluzioni che non sono mai arrivate, temporeggiando a più non posso per camuffare quello che ad oggi, con i licenziamenti sopraggiunti in questi giorni, appare come un *bluff.* Dalle chiacchiere della politica alle promesse della Whirlpool siamo presto giunti al tristissimo epilogo del licenziamento collettivo di ben 350 dipendenti della multinazionale appena terminato il blocco dei licenziamenti, termine che il Governo non ha voluto prorogare. La decisione della Whirlpool di chiudere il sito di Napoli il 31 dicembre 2020 per delocalizzare la produzione dove i salari risultano più bassi, nonostante un accordo con il Governo italiano e 50 milioni di euro di sovvenzioni pubbliche percepite dal 2014, rende drammatica la condizione degli operai che erano coinvolti direttamente nella produzione e quella di circa 1.000 lavoratori dell'indotto. Questo accade in concomitanza con la crisi causata da Covid-19, passata da emergenza sanitaria a emergenza sociale, che ha aggravato il quadro economico già precario di un territorio come quello campano, già fortemente depresso sul piano occupazionale. Nel frattempo dobbiamo ricordare che, mentre i Ministri trattavano con i vertici dell'azienda, nel bilancio del gruppo di fine 2018 erano già scritte a chiare lettere le intenzioni della Whirlpool in Europa e in Italia. In quel documento contabile, infatti, l'azienda, che aveva appena siglato l'accordo per tutti gli altri siti italiani, chiariva espressamente che avrebbe avviato forti azioni di recupero dei costi nell'area dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa. Ma veniamo ora agli errori odierni di questo Governo, che sapeva che, non prolungando il blocco dei licenziamenti, avrebbe innescato una crisi sociale senza precedenti, proprio in un momento di profonda crisi per tutta l'economia nazionale e mondiale. Come si può fare una cosa del genere? Davvero, colleghi, si è perso del tutto lo spirito della solidarietà e della salvaguardia sociale? Mi auguro che l'Esecutivo si impegni veramente al più presto per intervenire con misure straordinarie a favore di quei lavoratori, dal punto di vista non solo del sostegno economico,